Comunico che il 24 settembre 2020 l'ufficio elettorale regionale presso la corte d'appello di Venezia, a seguito dell'elezione suppletiva tenutasi il 20 e il 21 settembre 2020 nel collegio uninominale 09 della Regione Veneto, al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante per effetto del decesso del senatore Stefano Bertacco, ha proclamato eletto senatore della Repubblica il candidato Luca De Carlo. Comunico che, in data 25 settembre 2020, l'ufficio elettorale regionale presso la corte d'appello di Cagliari, a seguito dell'elezione suppletiva tenutasi il 20 e 21 settembre 2020 nel collegio uninominale 3 della Regione Sardegna, al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante per effetto del decesso della senatrice Vittoria Francesca Maria Bogo Deledda, ha proclamato eletto senatore della Repubblica il candidato Carlo Doria.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

per il prezioso contributo e per il lavoro che abbiamo svolto insieme nel difficile percorso di conversione del decreto-legge Considerando il difficile contesto economico, oltre che sociale, che coinvolge il nostro Paese e tenendo conto anche del difficile contesto epidemiologico che ha attraversato i nostri lavori (colgo l'occasione per augurare ai senatori una pronta guarigione), ritengo sia stato svolto un lavoro proficuo e anche la disponibilità al confronto con le opposizioni è risultata utile a qualificare la nostra iniziativa. Voglio ringraziare il presidente Pesco che insieme a noi ha condiviso questo difficile percorso. Insieme al senatore Errani abbiamo condiviso un'impostazione politica precisa nella conversione del decreto-legge; migliorare il testo, lavorando su quattro macro temi e costruendo su questi il confronto con le opposizioni e, senza emendamenti dei relatori, operare attraverso riformulazioni presentate da tutti i Gruppi parlamentari su emendamenti di iniziativa parlamentare dei diversi Gruppi. È stato così possibile migliorare il testo, favorendo in particolare una soluzione positiva per il lavoro fragile, interpretando correttamente importanti investimenti necessari nel settore turistico, in modo particolare sulle imprese in affitto e sul termalismo; risposte positive ed importanti anche nel pacchetto terremoto ed estensione dell'esenzione del canone occupazione

Quando il confronto avviene su una linea politica precisa, restituiamo anche alla parola politica la dignità che merita. Il confronto quindi ha qualificato e qualifica la credibilità del Parlamento

Come è evidente a tutti, il decreto-legge n. 104 non solo si colloca all'interno della strategia generale di risposta alla pandemia e di rilancio dell'economia varata dal Governo, ma costituisce anche il ponte verso la nuova programmazione europea. L'Italia cioè ha a disposizione non solo i 100 miliardi di indebitamento netto utilizzati per proteggere il lavoro, aiutare le imprese e favorire la ripartenza del nostro Paese, ma ha a disposizione la più grande, importante e straordinaria opportunità per progettare e programmare un nuovo sviluppo economico, collocare cioè lo Stato al centro di un'azione indispensabile per favorire una nuova economia. La riconversione in chiave ecologica dell'economia risulterà decisiva per determinare nuova occupazione e nuova crescita, così come l'impegno dello Stato nel processo di digitalizzazione del nostro territorio aprirà una fase nuova per il nostro Paese e per il nostro sistema economico. Abbiamo fatto tutto questo mettendo al primo posto il diritto alla salute. Promuovere la qualità del sistema sanitario e programmare i necessari investimenti per caratterizzare il nuovo volto della medicina territoriale non è utile solo per rispondere al primario diritto alla salute, ci consegna un nuovo significato del termine «pubblico». Lasciamo così nel passato la contrapposizione tra pubblico e privato, tra lo Stato e il mercato, tra il lavoro ed il capitale. Portiamo nel futuro una nuova funzione dello Stato e dell'intero sistema pubblico. Credo che si possa dire che potremo mettere fine ad un'inutile e strumentale contrapposizione politica verso tutto ciò che è pubblico e ricollocare il ruolo dello Stato dentro le dinamiche economiche.

alla digitalizzazione, all'università e alla ricerca, indispensabili per costruire una nuova agenda economica nel nostro Paese. Tutto questo avviene, Presidente, all'interno di dati e numeri che non possono lasciare alcun dubbio rispetto alla qualità della risposta che il nostro Paese ha dato e il nostro Governo ha individuato per attraversare la crisi. non è solo quello della qualità del lavoro del nostro sistema sanitario, che chiaramente ha dato prova di essere un sistema sanitario universale frutto del lavoro e dell'intelligenza del sistema pubblico più prezioso e più importante che, insieme alla scuola, abbiamo a disposizione. Sono i dati dell'Istat a confermare le misure importanti introdotte dal Governo, perché dopo un secondo trimestre molto negativo, il risultato del trimestre che va da maggio a luglio ci incoraggia verso una nuova ripartenza: per cento in valore assoluto sul PIL, più 11,5 in termini reali. Questo è il confronto rispetto al trimestre febbraio-aprile del 2020. Possiamo avere idee diverse, avremmo magari messo in campo mezzi, azioni e iniziative alternative tra le diverse forze politiche, ma non è corretto denunciare l'assenza di un progetto e la debolezza delle misure che abbiamo introdotto. tempi e modi diversi in stretta relazione con le dinamiche europee e con le scelte importanti che la Banca centrale europea ha compiuto nell'interesse dell'Europa. Insomma, abbiamo costruito questa risposta in stretta sintonia con un nuovo volto europeo. Non c'è campo né per il sovranismo, né per inutili polemiche all'interno delle nuove sfide economiche che abbiamo di fronte. muove sui 25 miliardi di indebitamento netto che il Parlamento ha autorizzato; 32 miliardi è il saldo netto da finanziare. Sono 100 miliardi di euro la risposta dell'Italia alla crisi pandemica, che rappresentano 6 punti percentuali di PIL, e altri 200 miliardi ovviamente di saldo netto da finanziare. Il decreto guarda oltre l'emergenza, spinge il Paese verso la ripresa delle produzioni e dell'occupazione.

12 in termini di saldo netto da finanziare che abbiamo utilizzato per rafforzare gli ammortizzatori sociali, rendendoli più selettivi, e per incentivare la ripresa dell'occupazione con sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato e per chi fa rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione. Per le aziende che hanno utilizzato gli ammortizzatori e non li richiederanno abbiamo previsto l'esonero dei contributi previdenziali a loro carico per i prossimi quattro mesi, entro il 31 Insomma, restituire centralità al lavoro, favorire la buona e la piena occupazione sono interventi utili che vanno al di là della crisi pandemica e restituiscono centralità e dignità alla straordinaria questione che il lavoro rappresenta. Ovviamente anche le imprese che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre vengono escluse dal versamento dei contributi previdenziali per sei mesi dall'assunzione. Insieme alla proroga della NASPI, sono misure sono misure molto importanti e qualificanti del nostro lavoro. stessa questione riguarda la filiera dell'economia: tre miliardi di euro. Sono interventi certamente più selettivi rispetto ai decreti precedenti, ma tendono ad affrontare le criticità dei sistemi economici più deboli, dal turismo all'agricoltura, alle piccole e medie imprese

Mi riferisco al necessario contributo che dobbiamo dare a sostegno dell'attività dei Comuni, perché la ripartenza avviene insieme ed è un pezzo importante del decreto Se a questo aggiungiamo gli 1,3 miliardi alla scuola, con assunzioni di personale e con adeguate strutture per programmare la ripartenza, credo che siamo in presenza di un provvedimento importante, utile a restituire centralità al nostro Paese, alla ricostruzione e alla ripartenza di un'economia che ha bisogno di restituire dignità e credibilità al lavoro e all'impresa. Le misure che abbiamo introdotto sono quindi funzionali alla ripartenza e sono un ponte verso la nuova programmazione europea. *(Applausi)*.

comunque la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

un lavoro che si è basato sostanzialmente sul concetto di provare a dare un ruolo al Parlamento; certo, non su tutto; certo non abbiamo cambiato la struttura del decreto-legge,

hanno lavorato insieme a noi per cercare delle risposte. Ripeto che non è tutto e non intendo in alcun modo rovesciare il ragionamento in relazione al rapporto tra maggioranza e opposizione, però un passo lo abbiamo fatto e io credo che questo sia molto importante. Su questioni sensibili, dal turismo, alle terme, ai lavoratori fragili, abbiamo raggiunto intese che hanno portato a riformulazioni comuni di tutti gli emendamenti. Da questo punto di vista io penso che sia la strada giusta: lo pensavo prima quando non ce l'abbiamo fatta, lo penso soprattutto per il futuro e in primo luogo per il *recovery

l'emergenza, la continuità con i provvedimenti precedenti per dare seguito e continuità a una serie di misure prettamente emergenziali (cassa integrazione, come ha già detto il collega Manca, non voglio consumare nemmeno i dieci minuti) e, allo stesso tempo, la prospettiva, cioè il bilancio e il *recovery fund.* questo sia un elemento importante che ci ha consentito di raggiungere anche alcuni sensibili orientamenti. È chiaro che la scommessa decisiva per l'Italia, non semplicemente per il Governo o per la maggioranza ma per il Paese, per tutti noi è come affronteremo la svolta che siamo obbligati a fare sul *recovery fund* e sul bilancio. A me sembra che siano sostanzialmente tre le grandi sfide: quella tecnologica con il 5G, ma anche la capacità di fare un piano vero sulle infrastrutture e, come ci suggeriscono le emergenze di queste ore, un piano vero e straordinario sulla manutenzione del territorio del nostro Paese. Si tratta di una grande priorità che ci può vedere insieme a lavorare, così come l'altra grande sfida, il *green new deal*, cioè la transizione ecologica dell'economia; una politica industriale che sia segnata profondamente da questo aspetto: la lotta alle vecchie e nuove disuguaglianze, magari pensando finalmente - come il Governo ha annunciato - a una riforma fiscale, non a interventi che rischiano di disallineare un sistema fiscale già profondamente disallineato, oppure rivedendo gli ammortizzatori sociali per dare loro una sistemazione complessiva. Bisogna trovare il modo di comprendere fino in fondo che non c'è semplicemente il lavoro dipendente, ma ci sono tante forme di lavoro, a partire da una parte significativa di lavoratori partite IVA che rischiano di essere le nuove povertà di questo Paese. necessari un salto di qualità, un dibattito vero che faremo nei prossimi giorni; cercheremo di impostarlo, ma questo decreto-legge si colloca tra l'emergenza e questa scelta. A tal proposito voglio sottolineare un aspetto un aspetto che tutti i Gruppi - maggioranza e opposizione - hanno evidenziato nella discussione in Commissione. C'è bisogno di un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione, nella struttura centrale e decentrata, di figure e competenze tecniche specifiche che portino avanti i progetti del *recovery plan*. Questa è un'emergenza assoluta che - rispondendo

per esempio, alla scelta sul turismo per quello che riguarda il credito d'imposta dal 30 al 50 per cento per gli affitti; il fondo per le terme. Stiamo parlando di settori che pagano un prezzo altissimo a causa della crisi Credo sia importante sottolineare la scelta sulla tassa per gli ambulanti e per i ristoranti. Questo rappresenta ossigeno

tutti i Gruppi in Commissione istruzione, o il 2 per mille per le associazioni culturali, il tentativo di disegnare alcune strade che dovranno essere riprese nella legge

un intervento robusto sui lavoratori fragili, perché è giusto. Parliamo dei lavoratori veramente fragili, quelli più a

Da questo punto di vista, essendo uno dei punti su cui tutti abbiamo raggiunto l'intesa, penso che ci distingua per l'attenzione e la cultura sociale che tutti i Gruppi - ho piacere di dirlo - hanno portato avanti. Voglio sottolineare, sul fronte

quest'ultimo riguardo abbiamo richiamato la necessità che il Ministero e le Regioni facciano un piano straordinario perché la salute mentale, anche a seguito dell'emergenza Covid, è un'emergenza nell'emergenza. Sappiamo che è uno dei servizi che più duramente ha pagato i tagli e credo che questo sia un punto importante.

molto significativa, ovvero il fondo per la stabilizzazione di chi è impegnato nei lavori di ricostruzione. Sarà necessaria, nel bilancio, una norma ulteriore per assicurare una risposta strategica, ma in col Governo abbiamo assunto un impegno politico, a cui si potrà dare una risposta definitiva. Vorrei poi sottolineare un altro elemento,

si è giunti ad un ordine del giorno, che impegna il Governo a dare seguito e continuità a questo fondo. Infine sulla scuola ci sono molto interventi e, anche in questo caso, sottolineo le cose nuove.

specifici o no. Sono poi state aumentate le risorse, per le Province e le città metropolitane, per la messa in sicurezza delle strade. Abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti, il quale, colleghi, il Parlamento ha detto la sua. Spero che, dopo questo passo, potremo continuare nel dibattito sul bilancio, ferme restando naturalmente le diverse posizioni, dei diversi Gruppi. Ringrazio ancora tutti i colleghi, che hanno lavorato con impegno a questa soluzione e ringrazio il Governo, che ha dimostrato una reale capacità di ascolto.

con serietà e con correttezza, anche grazie ai contributi che abbiamo dato noi, che siamo parte dell'opposizione. Il decreto-legge n. 104 del 2020, il cosiddetto decreto agosto, contiene delle misure che, come tutti sappiamo, sono a sostegno dell'economia e sono necessarie a seguito della pandemia, che ha coinvolto il Paese. Il documento, nella sua versione originale, è composto da 115 articoli e da oltre 100 pagine, che però non hanno molto a che fare con la precedente "madre di tutte le riforme" e cioè il decreto semplificazioni. Il decreto in esame utilizza gli ulteriori 25 miliardi di euro di scostamento di bilancio, che il Parlamento ha autorizzato con una votazione definitiva

Ci troviamo in presenza di un decreto-legge che, come abbiamo detto nel confronto avvenuto in Commissione, è l'esatta fotocopia dei decreti-legge precedenti: si interviene per tamponare l'emergenza immediata, come è giusto che sia, ma senza avere una vera prospettiva Il decreto agosto definisce misure che incidono per 28 miliardi di euro in termini di indebitamento netto. Si tratta di maggiori spese pari a 19,2 miliardi di euro, mentre le minori entrate sono pari a 8,7 miliardi. Le risorse reperite a copertura sono pari a 2,4 miliardi di euro di minori spese e maggiori entrate per soli 630 milioni. Il provvedimento agisce

su disposizioni finali (212 milioni). Accanto ad alcune misure positive, alcune delle quali apertamente ispirate da proposte dell'opposizione precedentemente bocciate dal Governo, non trovano spazio le esigenze di famiglie e imprese. Tra le misure necessarie, la prima è contenuta all'articolo 1, che proroga di ulteriori nove settimane la cassa integrazione Covid-19, da usufruire in un periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 Il datore di lavoro che chiede la proroga di ulteriori nove settimane è tenuto a versare un contributo straordinario, un'addizionale calcolata in base al fatturato del primo semestre, rispetto allo stesso periodo Per quanto riguarda il turismo, va sottolineato che siamo in presenza di uno dei settori più colpiti dall'emergenza. Questo disegno di legge poteva essere l'occasione per eliminare una misura che si è rivelata inutile, come il *bonus* vacanze: è stato evidente dall'estate appena trascorsa che il *bonus* non ha trovato apprezzamento, né presso i turisti, né presso le strutture ricettive; dei 2,4 miliardi di euro stanziati ad oggi è stato utilizzato solo l'8 per cento. appurato questo fallimento, sarebbe stato opportuno accogliere le richieste delle associazioni di settore, che auspicavano una revisione della misura sostituita con l'istituzione di un fondo *ad hoc* da destinare alle aziende in crisi.

Anche la scuola non è stata trattata a sufficienza. Nel decreto agosto è disposto un incremento di risorse per la scuola di appena 70 milioni di euro; si tratta di risorse che, pur sommandosi ai precedenti 300 milioni, rischiano di non essere sufficienti per avere un sereno anno scolastico. agosto resta parziale e pertanto non è sufficiente. Grava su di esso la necessità di un'ulteriore mole di decreti attuativi per rendere efficaci le misure, che altrimenti rischiano di rimanere solo sulla carta. carta. La Corte dei conti stima che la prima versione del decreto-legge, al netto degli emendamenti, richieda almeno 28 decreti attuativi. Nella maggior parte dei casi (19 di essi), non è prevista una data di scadenza per l'emanazione degli stessi. stessi. I decreti attuativi da emanare vanno ad accodarsi ad altri mai emanati e facenti capo agli altri decreti-legge convertiti in legge nei mesi scorsi, da quando è scoppiata l'emergenza. In totale, su 252 decreti attuativi da emanare, ne mancano all'appello Tutto questo si traduce in risorse bloccate. In definitiva, in questo provvedimento manca l'immediatezza e si perde tutto nei meandri della burocrazia.

Mi riferisco, in particolare, a quelle disposte dall'articolo 11 «Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di Taranto», che autorizzano l'assunzione di 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, con un costo di circa 13 milioni di euro che è andata da poco al voto. Un'altra misura del ministro Franceschini riguarda una dotazione di 4 milioni di euro per il 2020 e 16 milioni di euro per il 2021 per incarichi di collaborazione fino a 40.000 euro ciascuno, per un totale di ben 500 collaborazioni.

in esame mancano, in qualsiasi contesto, interventi per garantire investimenti infrastrutturali, liquidità alle imprese e sostegni concreti alle famiglie. Il mantra del Governo è rinviare: ai tempi del decreto cura Italia le proposte di rilancio presentate dalla minoranza venivano bocciate, con la promessa di inserirle nel cosiddetto decreto aprile, poi diventato decreto maggio e, infine, decreto rilancio. Durante la discussione del decreto rilancio ci siamo sentiti rinviare alcune proposte al decreto agosto. Oggi il ritornello cambia ancora una volta e ci sentiamo dire che gli interventi strutturali saranno fatti con i fondi europei del *recovery plan.*

perché la Nazione è stanca e non saranno certo i decreti adottati in questi mesi a salvare il nostro Paese.

vorrei iniziare con un *mix* di note, alcune belle, alcune comiche, alcune serie, anzi serissime. È chiaro che siamo all'abuso della fiducia.

Il Mose funziona. Ripeto, nonostante anni di contestazione, il Mose funziona e questa è una bella notizia. L'altra bella notizia è che Trump sta meglio e se vincerà, come io spero, andrà a fondo su certe questioni che riguardano anche l'Italia.

Penso che non si possa tergiversare e che il Piemonte, in particolare nelle province di Cuneo, di Biella e di Vercelli, richieda investimenti pronti e senza tante complicazioni burocratiche. Esamino ora alcuni articoli a mio giudizio interessanti. «Strada sicura» conferma il contingente delle Forze armate che presta servizio nei punti nevralgici fino al 15 ottobre Penso che il maxiemendamento in preparazione debba correggere la data di scadenza e apporre il «15 ottobre 2021»; è un suggerimento al Governo e alla maggioranza per non perdere tempo con altri decreti. altri decreti. L'articolo 39 prevede la rendicontazione dei contributi ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, a ristoro delle mancate entrate e delle maggiori spese per il Covid.

e 3: una volta che il Governo ha dato il ristoro degli importi non incassati e delle maggiori spese, finisce lì; la rendicontazione al 15 aprile in assenza di dati certi è una complicazione unica e difficilissima. previsti 300 milioni a ristoro parziale dell'imposta di soggiorno, con un decreto ministeriale per la ripartizione.

2021-2023, per i ponti. Di ponti avevo già parlato in altri interventi e le alluvioni dimostrano che sono un discorso quanto mai attuale e delicato.

riguarda la partecipazione diretta e indiretta al capitale delle imprese.

siamo da capo, secondo me sono soldi buttati nel pozzo.

l'articolo 87 siamo all'apoteosi: costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica; si affitta la compagnia che sta per fallire, ma non si farà fallire: con un piano industriale, che è pubblico, sono stati stanziati altri 3 miliardi di euro, assieme alle centinaia di milioni dei precedenti decreti. Credo che questo sia veramente uno sbaglio storico che pagheremo caro con figuracce internazionali, con disservizi e risultati

di ascoltare i suggerimenti di alcuni studiosi e giornalisti *super partes* - o quasi - che chiedono di fare una norma che renda facoltativi gli ammortamenti nei bilanci della società per il 2020. Credo sia possibile per un anno non fare gli ammortamenti in un bilancio e presentare un bilancio attivo, o vicino all'attivo, in un momento di difficoltà. A mio avviso, e concludo, non c'è una strategia di insieme: c'è un po' di tutto, buttato lì. Vediamo cosa succede, ma i sussidi a pioggia non portano vantaggi Bisogna favorire gli investimenti, come si è tentato di fare - e sottolineo «tentato» - nel decreto semplificazione, ma devono partire. Non basta rinviare le tasse: bisogna prevedere l'abolizione di alcune tasse

Signor Presidente, membri del Governo, è ormai una triste realtà quella dei provvedimenti di questo Esecutivo, che denotano un immobilismo surreale, che diventa oggi ancora più lampante alla luce della grave situazione che il nostro Paese sta vivendo per l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest, compromettendo la vita dei cittadini, la viabilità, i territori, gli edifici privati, le imprese e le opere pubbliche. L'alluvione di tre giorni fa, le piogge incessanti, gli alvei dei fiumi pieni di detriti e ostruiti da ghiaia e tronchi di alberi hanno messo in ginocchio il Nord-Ovest del Paese. Il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria stanno contando i danni. Da una prima sommaria stima effettuata oggi dalla Coldiretti, i danni per gli effetti devastanti del maltempo solo su agricoltura e imprese si parla di altrettanti danni per le opere pubbliche. Migliaia di cittadini sono rimasti senza elettricità, telefono e gas, con intere frazioni e comunità isolate. Il bilancio provvisorio parla di almeno otto morti e di un disperso. È una situazione complicatissima, collegamenti nazionali e internazionali strategici completamente fuori uso, tra cui la strada statale del Colle di Tenda e il relativo tunnel, che collega l'Italia alla Francia, un'arteria internazionale fondamentale per il sud del Piemonte. La situazione è drammatica ovunque,

In queste ore i sindaci, gli amministratori locali, gli uomini della Protezione civile, i volontari, i privati, centinaia di persone si stanno dando da fare e sono a lavoro per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori. *(Applausi)*.

telefonando direttamente al Governatore del Piemonte ieri mattina. Il presidente del Consiglio Conte, invece, si è preso un po' più di tempo: è riuscito a telefonargli oggi a mezzogiorno,

fronte ad una fragilità del Nord-Ovest già evidenziata - nel 1994, quando ci fu l'alluvione con decine di morti, e nel 2016 la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, ha cercato di porre rimedio già in questo provvedimento, nel decreto agosto, attraverso un emendamento sul dissesto idrogeologico, con l'istituzione di un fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni, con una dotazione da 100 milioni di euro che, tuttavia, non è stato approvato - lo sanno bene i nostri colleghi della Commissione bilancio - ma accolto come ordine del giorno.

dal titolo «I soldi contro il dissesto ci sono, ma i Comuni non sanno come spenderli». Siamo alla follia di un Governo allo sbando, che fa lo scaricabarile sui sindaci.

Signor ministro Costa, glielo diciamo da quest'Aula: i decreti attuativi li fanno il Ministro e i Ministeri, non li fanno i sindaci, i consiglieri regionali o le Regioni. Si assuma le sue responsabilità, che sono gravissime! Tiri fuori la dignità e la professionalità e la applichi al Ministero, invece di andare ad incolpare delle persone che non hanno nessuna colpa in questo caso. Ci vuole, da subito, un decreto che dichiari lo stato di calamità e di emergenza immediato con risorse certe e nomini i Presidenti di Regione, i nostri governatori, come commissari, al fine di accelerare le procedure per ripristinare lo stato dei fatti. Ci sono strade internazionali completamente impraticabili in questo momento. Su questo, sulla pulizia degli alvei dei fiumi e su tutto quello che riguarda la sistemazione dei torrenti, ricordo al Ministro e al Governo che abbiamo depositato un provvedimento nell'aprile del 2018, a prima firma del nostro collega senatore Paolo Arrigoni ma lo abbiamo firmato tutti noi membri del Gruppo Lega-Salvini Premier, ed è un disegno di legge nel quale si dà la responsabilità ai sindaci e ai governatori di stabilire le procedure d'urgenza per la pulizia degli alvei, una semplificazione. Questo provvedimento è fermo perché il Presidente della Commissione ambiente del Senato indossa la maglia

Se vogliamo, Presidente, salvare il Nord-Ovest da questo dramma, ci vogliono risposte certe, immediate e concrete, come fece il nostro sottosegretario Vannia Gava, che nel 2019 per il dissesto idrogeologico finanziò i Comuni con 315 milioni di euro veri, non parole, non farfalle, ma soldi veri. *(Applausi).* Rivolgo un invito finale al Presidente del Consiglio e al ministro Costa

Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, intendo soffermarmi in particolare su un segmento normativo di questo importante pacchetto, pacchetto, che riguarda il rafforzamento e l'ampliamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne, un argomento di grande importanza non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale e culturale, anche perché riguarda un ambito vastissimo del territorio nazionale. Le aree interne coprono il 60 per cento dell'intero territorio nazionale, il 52 per cento degli 8.000 Comuni italiani

e 28-*bis* del decreto. Le aree interne hanno subito negli ultimi tempi uno spopolamento veramente pauroso, hanno alimentato in misura preponderante il deflusso demografico dal Mezzogiorno, che registra negli ultimi dieci anni la perdita di un milione di abitanti e di 200.000 laureati, per la cui formazione lo Stato ha impiegato 34 miliardi di euro. Questo

a quel grido di dolore - lo dico senza enfasi - che nasce da decenni di solitudine in cui hanno vissuto le aree interne - attenzione, non solo del Sud, ma anche del Nord anche del Nord - che nel loro complesso formano, come dicevo poc'anzi, oltre la metà dell'intero territorio nazionale. Quali sono le ragioni sono sotto gli occhi di tutti: l'assenza dei servizi. Basti dire che un indicatore molto significativo riguarda il Servizio sanitario. I centri di montagna e di collina lontani dai poli del Servizio sanitario

Ancora, la banda larga serve per il 30 per cento le famiglie italiane in generale; per il 70 per cento le famiglie italiane sono prive della banda larga e la parte preponderante di questo 70 per cento è nelle aree interne

nella misura in cui inverte con decisione una tendenza alla dimenticanza, all'abbandono, alla condanna e alla solitudine. L'articolo 28 aumenta considerevolmente la dotazione finanziaria sia

relativo decreto interministeriale non costituisce, come dicono i tedeschi, una *Blankovollmacht*, una procura in bianco, ma fissa criteri molto precisi che sono lodevoli e apprezzabili: la deroga alla chiusura degli istituti scolastici nelle zone montane, insulari e periferiche e l'introduzione di forme di premialità per i docenti

perché contrasta la dispersione scolastica e l'abbandono del servizio scolastico. Concludo, Presidente, con riferimento ad un'altra questione molto importante, un altro aspetto che deve essere sottolineato.

e alla strategia associativa necessarie per contrastare gli *handicap* che nascono dall'assenza di fenomeni di urbanesimo e dalla polverizzazione urbanistica sul territorio. I piccoli Comuni non sono in grado di svolgere efficacemente i vari servizi pubblici se non attraverso una strategia associativa. Questo è scontato nell'ambito di questa strategia associativa, è estremamente importante e necessario mettere in rete i valori i valori culturali del territorio. Mi riferisco alle risorse paleontologiche, archeologiche e delle arti figurative. I piccoli Comuni hanno una presenza disseminata di questi attrattori turistico-culturali che di per sé, isolatamente, non hanno *appeal*, un'efficacia rilevante, ma con la messa in rete si crea un fenomeno di sinergismo che richiede necessariamente una strategia associativa. I fondi previsti dall'articolo 28 devono allora essere diretti soprattutto a sostenere e incentivare questa strategia associativa. Un'ultima raccomandazione al Governo, se mi è consentito, è quella di fare presto. Presidente, è in corso una lotta contro il tempo; secondo l'Istat, se non si provvede a invertire la tendenza l'80-85 per

mette in condizione i cittadini di non perdere la fiducia, perché una cosa è vedere le realizzazioni concrete, altra cosa è vedere promesse astratte che non si non si traducono in acquisizioni reali.

il provvedimento che stiamo discutendo e che voteremo, il decreto agosto, stiamo avendo la conferma del virus costituzionale diffuso dal Governo Conte-*bis*, virus che sta colpendo una delle principali istituzioni dello Stato: il Parlamento. Le poche risorse destinate all'attività emendativa riservata al Senato sono la riprova della scarsa considerazione nei confronti dei parlamentari eletti dal popolo, ricordando così il metodo recidivo delle continue fiducie, sommate ai ritardi e ai problemi di accordi di maggioranza, che pregiudicano una tempistica ragionevole per poter valutare i provvedimenti da entrambi i rami del Parlamento, di fatto esautorando i parlamentari dal loro ruolo. Ne è un esempio il recente risultato elettorale delle elezioni del Consiglio regionale veneto, una Caporetto che ha travolto alcuni partiti. Questo è indice di una parte del tessuto politico e di rappresentanti politici slegati dalla realtà, a livello parlamentare e a livello regionale, indaffarati a demonizzare la politica amministrativa lungimirante del governatore Luca Zaia, frutto di un continuo confronto col territorio, con il tessuto sociale, le aziende, gli imprenditori, gli artigiani e gli agricoltori. Se continuerete a perseverare a partorire provvedimenti senza l'ascolto del territorio, darete il colpo di grazia a questo Paese, già provato anche dagli effetti economici, oltre che sanitari, della pandemia. Quando tornerete a casa sarà già tardi. Speriamo succeda il più presto possibile. *(Applausi)*. a cosa l'attuale Governo sta solo pensando (ripeto, sta solo pensando ma non è nemmeno da pensare). È un peccato avere questi pensieri: la riduzione di orario di un ristorante alle ore 23. Concentrare le stesse persone in un orario ridotto è improvvisazione, incapacità e malafede. Come si fa a non capire che così i rischi aumentano? Anche in questi giorni sono stato in contatto con persone e realtà del territorio nazionale, e non parlo del Veneto ma del Sud del Paese. Anche in Sicilia la lamentela e la constatazione è che la semplificazione è lontana anni luce da quella che sarebbe una sburocratizzazione necessaria e fondamentale per il nostro Paese. Serve qualcosa di diverso. Con il decreto agosto viene confermata la disorganicità dei provvedimenti: soldi calati con marchette che non porteranno a una crescita concreta. Gli amici del Sud confermano che serve *in primis* una rivoluzione culturale e amministrativa; dare loro soldi senza un'opportuna progettualità non porterà a niente. L'attività emendativa della Lega è stata ridotta all'osso e che poi non si venga a dire che non abbiamo collaborato. rivolta un'attenzione verso il Sud ma senza discriminare altre parti del Paese. Ricordatevi che il Nord vuole tornare a essere protagonista, certo non senza il Sud. Il Nord deve essere la locomotiva ma sicuramente le altre regioni devono essere vagoni del treno dello sviluppo. Inoltre, a mio modo di vedere, il sistema Italia vuole tornare a essere grande per farlo si deve iniziare valorizzando maggiormente il mondo dell'agricoltura nella giusta maniera, come di seguito indicherò. Occorre internazionalizzare il *made in Italy*. I prodotti agricoli, i manufatti, tutte le eccellenze che fuoriescono dal mondo agricolo italiano devono essere portate sul mercato estero per il tramite dei consolati e delle ambasciate, che devono aprire sezioni al loro interno proprio per appoggiare, supportare, essere di ausilio e favorire le imprese italiane già presenti in quei territori o che vogliono entrarvi. Il Ministero degli affari esteri deve diventare, tramite le sue propaggini presso gli Stati esteri, promotore di sviluppo economico a partire dall'agricoltura. L'internazionalizzazione del *made in Italy* non deve essere aiutata solo sotto l'aspetto economico, finanziario e fiscale ma in modo diretto nei territori esteri dove deve il più possibile diffondersi. Ci servono investimenti subito per l'irrigazione e per la bonifica a seguito dei cambiamenti climatici che ci impongono in particolare di concentrare una grande attenzione sulla bonifica, garante del corretto deflusso delle acque.

Parlo di quello che io da sindaco - al terzo mandato - ho visto con i miei occhi e toccato con le mie mani all'interno di un consiglio di amministrazione di un consorzio di bonifica, quello veronese, dove ero rappresentante dei sindaci. La progettualità non manca. I sindaci sanno benissimo cosa vogliono e a fianco hanno degli enti di natura

perché sanno portare avanti la progettualità. Quest'ultima è vista in prima persona dalle amministrazioni, dai Comuni e dai sindaci, ma sicuramente sulla progettualità l'ANBI, a livello nazionale, non farà mancare Gli investimenti, quindi, servono per la cura e contro l'abbandono del territorio. Troppi agricoltori lasciano le zone di montagna per lo scarso reddito o perché questo Governo, con il ministro Costa e il ministro Bellanova, non vogliono affrontare il problema dei danni da animali selvatici. anche sulle opere idrauliche, che si stanno verificando in molti territori italiani e che posso, come ho già detto prima, personalmente toccare con mano visto che il mio territorio della Bassa Veronese non ne risulta esente. Ci servono poi finanziamenti subito per la meccanizzazione agricola. Abbiamo un parco macchine vecchio, troppi sono gli incidenti sul lavoro in agricoltura e ce lo dice anche l'INAIL. Non si risolve il problema importando 600.000 immigrati. Alla nostra agricoltura servono nuovi macchinari, nuove tecnologie, non ci servono immigrati da mantenere. inoltre interventi fin da subito per aiutare il settore florovivaistico messo in ginocchio dal *lockdown*, così pure per il settore agrituristico. Quest'anno non sono arrivati i turisti stranieri e quindi all'agricoltura è mancata gran parte della domanda del settore della ristorazione sia per l'agricoltura, che per l'allevamento e il settore caseario. Per queste motivazioni spero che la parte che riguarda il coinvolgimento dei Gruppi di minoranza sia sempre più proficua perché in questo decreto-legge non c'è stato per nulla. Mettete una mano sul cuore e sulla coscienza e sappiate coinvolgere di più i parlamentari di opposizione.

oggi potrei iniziare con facilità citando delle realtà economiche e sociali che certamente sono ben più vicine a me. Potrei ricordarvi, usando le parole del presidente della Confindustria, che non vorremmo morire nel regno del Sussidistan. Potrei ricordarvi, sempre riferendomi al presidente Bonomi di Confindustria, che che il decreto agosto prevede interventi frammentati e senza visione. Potrei, quindi, esordire, riferendomi alla parola di coloro che rappresentano il mondo dell'impresa in Italia. E invece no.

dicendo che bisogna uscire dalla logica emergenziale e che bisogna finalmente avviare la ripresa. Non vi cito le parole del mondo economico, degli imprenditori e dei padroni, come molti di voi li definiscono, ma quelle usate in queste ore - non avrei mai pensato di farlo - da colui che, forse, è il più lontano dalla mia visione politica, ovvero dal segretario della CGIL. Perfino dalla CGIL vi fate richiamare alla concretezza, alla necessità di venir meno alla logica emergenziale dei sussidi. Stiamo parlando del quinto decreto Covid: dopo il cura Italia, il liquidità, il rilancio e il semplificazioni, adesso abbiamo anche il decreto agosto perché ovviamente non avevate più nomi credibili per poterlo nominare e vi siete semplicemente rifatti al mese della sua stesura. Colleghi, come tutti gli altri decreti-legge, è perfettamente consequenziale: abbiamo un ulteriore decreto-legge che è esattamente la continuazione logica di pensiero operativa della vostra inconsistenza pratica. Si tratta pieno di decreti attuativi da realizzare. Vorrei ricordarvi che Openpolis pochi giorni fa ha quantificato in oltre il 70 per cento i decreti attuativi non realizzati per dare efficacia ed efficienza ai vostri provvedimenti. Vorrei ricordarvi i fallimenti ai quali siete andati incontro e state continuamente andando incontro con i *bonus*.

Ricordo il *bonus* monopattino, l'ennesima marchetta a qualche realtà imprenditoriale asiatica cinese

Vogliamo procedere con un'altra presa in giro delle nostre imprese. Ci ricordiamo tutti quando avete introdotto il credito sanificazioni. Era una delle poche cose giuste che ho letto nei vostri decreti. Quel credito di imposta che doveva essere del 60 grazie al fatto che non sapete nemmeno quantificare i soldi che servono e che vengono impiegati e quelli che non servono e non vengono utilizzati, come ho detto prima, e grazie

Proseguendo, quali sono le misure per la ripresa, qual è il coraggio che non c'è stato nel decreto semplificazioni? Potete interloquire tranquillamente con dirigenti dei settori appalti pubblici di qualunque colore politico - lo sottolineo - e vi diranno che non avete fatto nulla per semplificare il mondo degli appalti, quindi nemmeno in un'emergenza come questa, nemmeno in un momento straordinario come questo, siete stati capaci di dare risposte a coloro che non riescono a far partire gli appalti in questo Paese. Siete proni a una logica giustizialista e burocratica; siete incapaci, finanche in emergenza, di dare risposte al Paese.

fra poche ore, 9 milioni di cartelle esattoriali penderanno addosso ai nostri imprenditori, alle nostre piccole e medie imprese, alle nostre famiglie. Non vi siete ricordati di questo,

dei soldi che avete regalato come mance e mancette: magari i 4 milioni che avete previsto negli emendamenti al provvedimento in esame e che avete assommato ai 4 milioni che già avete regalato nel decreto rilancio

non voglio dire che non siano finalità anche lecite, al di là del merito, ma non erano certo queste le finalità di un decreto-legge che doveva servire a rilanciare il nostro Paese: queste sono mance che la politica che sostiene il Governo sta vergognosamente elargendo alle spalle degli italiani. Pertanto, cercando di sintetizzare perché il tempo non è tanto, vorrei chiedere a voi cosa avete pensato di fare per i professionisti.

far riferimento all'ecobonus. Anche in questo caso state vanificando una misura di primaria importanza. L'ordine degli ingegneri di Torino ha scritto a tutti i membri del Governo per caratterizzare le incapacità operative alle quali li state sottoponendo, per sintetizzare i problemi che hanno

i problemi del credito che la precedente riforma della scorsa legislatura ha evidenziato, rovinando completamente il credito del territorio. del credito che vede oggi soccombere le piccole banche e che vedrà soccombere le nostre aziende e la capacità di credito delle banche per il fatto che al termine della moratoria dovremo andare a rivedere i *rating*. In questo modo i nostri istituti di credito non avranno più capacità

sui problemi della proprietà edilizia: sfratti per i quali non è stato previsto alcun indennizzo per i proprietari che stanno soffrendo. Ricordo i canoni di locazione non pagati per i quali soffrendo. Ricordo i canoni di locazione non pagati per i quali i proprietari devono, però, continuare a pagare le tasse, perché vale il principio di competenza. Cosa state facendo per questi proprietari immobiliari che non riescono ma devono pagare le imposte anche sui canoni che non sono stati pagati?

devo essere d'accordo con coloro che ritengono questo decreto-legge l'ennesima dimostrazione di una politica propagandistica e incapace di dare risposte ai cittadini e agli imprenditori di questo Paese.

Prima di fare una valutazione completa su quella parte, mi preme una riflessione su quanto è stato detto poc'anzi, che investe anche le competenze del Ministero di riferimento della mia Commissione. Mi riferisco in particolare ai fatti tragici avvenuti recentemente in Piemonte e in Liguria. Penso che, rispetto alle parole che ho sentito, non serva fare leva sulle sciagure delle persone per evidenziare il proprio pensiero, la propria richiesta, la propria proposta. Sono nelle cose la vicinanza, il sostegno, la solidarietà verso quei residenti che sono stati provati per rimettere in funzione un territorio così duramente colpito. Quindi, non serve, ogni volta che accade qualcosa, rivendicare una primazia, così come ho ascoltato in quest'Aula, come se gli altri avessero maggiormente a cuore le difficoltà del nostro Paese. È una sciocchezza, è sempre stata tale e continuerà a esserlo perché, come è noto, quanto serve per ripristinare quei luoghi sarà fatto. Non vi siano dubbi:

Anzi, il paradosso assoluto è che, da una parte, ci sono le parole; dall'altra, ci sono i fatti. Nell'ambito di questo decreto-legge anticipiamo 3 miliardi di euro dal 2030 al 2020-2021 proprio per la messa in sicurezza del territorio. Scommettiamo che quel collega tra poco voterà contro il decreto-legge agosto? Scommettiamo che voterà contro il decreto-legge agosto all'interno del quale 600 milioni di euro sono destinati ai ponti, compreso quello che alcuni sindaci sono andati a inaugurare poco prima che cadesse? Ecco la propaganda. Saprebbe dirmi quel collega qual è la procedura diversa che è stata utilizzata quando governava lui, quando il Veneto è stato colpito dalla tempesta Vaia nell'ottobre 2018? La stessa identica che c'è sempre stata per tutte le tragedie di questo tipo e che ci sarà anche per quella che ha colpito ahinoi - il Piemonte e la Liguria. Quindi non serve quel tipo di comportamento: gli italiani sanno bene come funziona nel nostro Paese. Cerchiamo di accelerare e di rendere le procedure sempre più semplici, ma nessun italiano, rispetto a quelle tragedie, sarà lasciato indietro. il relatore Manca ha detto che all'interno del decreto-legge in esame ci sono i prodromi e gli indirizzi chiari della nuova programmazione europea. Ha perfettamente ragione: quello è il vero tema, sul quale ci confronteremo a breve, a partire dalle linee guida, per arrivare poi alla pianificazione più dettagliata. All'interno del decreto-legge in esame vi sono degli indirizzi chiari del nostro progetto politico, a sostegno di tutte le difficoltà, che sono state determinate, ahinoi, dalla pandemia. Vi sono quindi sostegni concreti per i lavoratori marittimi, per il settore aereo e per il trasporto ferroviario locale e regionale. Vi sono ingentissime risorse per gli enti locali: in precedenza ho fatto riferimento alla misura dell'anticipo, dal 2030 al 2034 a quest'anno e all'anno prossimo, di circa 3 miliardi di euro, ma vi sono altri fondi per le opere pubbliche di efficientamento energetico, per lo sviluppo territoriale sostenibile, per la messa in sicurezza dei ponti, a cui ho fatto già riferimento, già riferimento, e per la progettazione di opere pubbliche da parte degli enti locali. Si tratta di un volume di risorse, ahinoi dettate dall'emergenza, ma che, con assoluta chiarezza, fanno trasparire la nostra volontà politica di sostenere ogni azione delle pubbliche amministrazioni, a sostegno delle difficoltà delle persone e, in questo caso, in alcuni aspetti, del nostro territorio nazionale. Abbiamo un'attenzione dedicata, attraverso il programma pluriennale, a potenziare tutti gli investimenti sulla sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici. Che dire poi del fondo a sostegno di tutte le politiche in favore della Pianura padana? C'è qui uno specifico riferimento alla promozione di strategie, che puntano sì alla migliore infrastrutturazione, ma anche alla migliore qualità qualità dell'aria. C'è poi il sostegno per gli esercenti del trasporto di linea di persone, effettuati su strada mediante gli autobus. Abbiamo considerato di tutto, dal trasporto marittimo dei passeggeri, con 50 milioni di euro, all'autotrasporto dei passeggeri su strada,

il termine per la scadenza della concessione, che è scaduta il 30 aprile 2014. Quell'emendamento era più completo ed è stato considerato in parte inammissibile: lo valuteremo nelle prossime settimane, in occasione dei prossimi provvedimenti. Quell'operazione blocca blocca una concessione autostradale, che vale circa 4,5 miliardi di euro di investimenti sui territori interessati da quell'infrastruttura. Spero sia l'ultima volta che sarà rinnovata la proroga: lo dico con assoluta chiarezza. Ritengo che molte delle cose dette, che impediscono il rinnovo della concessione, non siano vere, come quella per cui l'Europa dovrebbe decidere, se anche restassero i privati, che sarebbero affidamenti *in house* o altre cose. Auspico resilienza e responsabilità da parte di tutte le forze politiche, affinché sin dalla prossima legge di bilancio ci possa essere una soluzione definitiva. Il Partito Democratico

delle ferrovie interregionali, che vanno sulla tratta ferroviaria da Bologna al Brennero e quelle da Venezia a Trieste, passando per Udine, per quanto riguarda la Regione Friuli. È un mio emendamento sulla concessione in gestione delle ferrovie interregionali. Non ho avuto bisogno di essere a favore del *referendum* sull'autonomia: si può fare, questo è il principio della sussidiarietà. Non abbiamo bisogno di gente che ci ripete che ci ripete che le Regioni dovrebbero gestire in autonomia; stiamo dimostrando, come Partito Democratico, che il nostro principio della sussidiarietà passa attraverso le leggi in vigore. Non c'è bisogno di propaganda, le cose si possono fare e questo lo dimostra.

in quelle località. Ci sarebbe molto da dire anche sull'Autorità che abbiamo istituito per la laguna di Venezia, rispetto alla quale il segnale positivo di sabato sul funzionamento del Mose, finalmente, dopo tante ruberie e dopo tanti contrasti, ha dato un motivo di orgoglio al nostro Paese. Speriamo che continui a funzionare; quantomeno abbiamo tacitato la bocca a coloro che hanno detto che quell'opera non avrebbe funzionato. Signor Presidente, concludo davvero e la ringrazio per la sua cortesia. Ho iniziato dicendo che aveva ragione il relatore Manca: è vero, perché questo provvedimento ci dispone in quella direzione; questo impegno ci dispone al dispiegamento delle ingenti risorse che l'Europa ci ha concesso. Stiamo dimostrando di saperlo fare e lo faremo per il bene dell'Italia.

e lei lo sa. Questo è uno dei punti più importanti del nostro dibattito in questo momento: il Governo non ascolta. Non ascolta quando siamo in Aula e non ascolta nemmeno quando parliamo in altri luoghi e in altre circostanze.

già questo dimostra un ritardo tra la pianificazione degli interventi che è stata fatta oltre due mesi fa e l'evoluzione della situazione che stiamo vivendo in questo momento. Forse due mesi fa venivamo dalla speranza che una fase della pandemia si fosse in qualche modo conclusa; ci presentavamo all'opinione pubblica, anche a livello europeo, come il Paese che prima, più e meglio aveva saputo gestire la situazione. Disgraziatamente, il concatenarsi degli eventi ci dimostra come, anche in Italia, in questo momento ci sia una ripresa della pandemia, con un *trend* in crescita - ringraziando Iddio inferiore a quello che succede in Francia e in Spagna, i Paesi a noi vicini, ma certamente un *trend* in crescita - che coinvolge l'Italia in una progressione continua. Quali sono le ragioni di questo *trend*, di questa sorta di pandemia sanitaria legata al virus, che però trascina con sé altre due questioni, che in questo momento stanno appesantendo notevolmente il nostro Paese? Una è quella economica: molti dei colleghi intervenuti hanno fatto riferimento a tale questione, che il Governo finora ha gestito con mentalità prevalentemente assistenziale; non l'ha certamente gestita con l'intenzione, con l'impegno e con le decisioni necessarie a rimettere in moto l'economia. Se c'è un anello debole in tutto questo sistema è proprio la povertà culturale, la povertà strutturale delle decisioni che avrebbero dovuto dare ossigeno in tempo reale alle aziende.

luogo, probabilmente remunerati non tanto quanto si potrebbe avere con il reddito di cittadinanza. Tutte le sere c'è un'azienda che ci racconta la difficoltà che ha a trovare manodopera.

e probabilmente una sorta di prosciugamento (a meno che non ci vorremo investire la maggior parte dei fondi del *recovery fund,* quando arriverà) di quella che in un certo senso è l'indennità di disoccupazione, cioè la cassa di disoccupazione.

di diventare parolaia, buona da spendere in televisione e per fare degli annunci, ma del tutto vana quando si tiene in conto che mancano i famosi 181 decreti attuativi

In questa logica, che è la sagra dell'incompetenza strutturale, stiamo condannando il Paese anche a un'altra operazione composita che riguarda il mondo della scuola. scuola. Ci vuole davvero coraggio ad andare in televisione a dire che per la scuola va tutto bene. Bisogna sentire gli insegnanti

Voglio dire una cosa: noi ci auguriamo di avere un Governo, non dico illuminato e competente, non dico orientato a fare il suo lavoro e a scrivere i suoi decreti attuativi; non dico questo, ma che almeno abbia l'umiltà, quando è in Aula, di ascoltare i colleghi dell'opposizione. Signor Presidente, dovremmo dire che non c'è due senza tre, visto che ci sono altri 25 miliardi di scostamento che noi responsabilmente abbiamo votato e che portano il totale ad oltre 100 miliardi. Purtroppo, ci ascoltate quando si tratta di votare lo scostamento, ma non ci ascoltate praticamente mai quando si tratta di decidere come impiegare le risorse, se non per quegli argomenti che sono talmente evidenti che non li si può negare. Peccato allora che il re - e anche il "Conte", mi permetto di dire - sia nudo e il *bazooka* sia scarico. Oggi persino il Presidente del Senato ha richiamato alla necessità di dire le cose come stanno e quello che serve fare.

dalla situazione che si è creata in numerose Regioni per il disastro causato dai nubifragi e dal maltempo. Mi dispiace, collega D'Arienzo, ma serve ricordarlo in quest'Aula; non permette di risolvere, ma serve ricordarlo ed è doveroso per non essere complici. ci ha fatto un elenco di tutto quello che non serve, puntuale ma non condivisibile; io aggiungo una cosa che non serve fare: è inutile dire quanto si stanzierà nel 2031 e non dire perché non si è fatto qualcosa l'anno passato, perché non si sta facendo qualcosa quest'anno e perché non si accelereranno gli investimenti in maniera più consistente di quanto è stato fatto con questo decreto-legge. Si chiedeva provocatoriamente: «che cosa avreste fatto voi?». Sicuramente avremmo approvato oramai, se non fossimo stati rallentati da una forza politica ben precisa - e mi riferisco ai 5 Stelle - quel disegno di legge che il 4 aprile del 2018, insieme al collega Arrigoni, come Lega abbiamo depositato per semplificare la pulizia dell'alveo dei fiumi e dei torrenti. Non è la prima volta, purtroppo, che lo ricordiamo. Ecco, quello sarebbe stato possibile fare se quel disegno di legge fosse stato calendarizzato e approvato. Allora facciamolo ora. Non significa approvarlo alla lettera, per come è stato depositato, ma si può prendere una buona volta un impegno corale - qualche volta l'abbiamo fatto - e unanime in quest'Assemblea? Si può calendarizzare in Commissione ambiente quel disegno di legge, abbinargliene magari altri ed arrivare a una pronta approvazione, perché sia questa veramente l'ultima volta Ci sono altri emendamenti che abbiamo presentato, non provocatori, che cercavano di completare, magari anche con qualche spunto valido. Perché trovare all'articolo 11 del decreto-legge in discussione un importante sacrosanto intervento per l'arsenale di Taranto e negarlo all'arsenale di La Spezia? C'è qualcosa di diverso? *(Applausi).* Se è ammissibile intervenire, giustamente, per accelerare le assunzioni per l'arsenale

proprio per l'assenza delle assunzioni? Ricordo che questa era l'impegno che aveva preso il ministro Guerini non con noi, non con l'opposizione, ma ad esempio con l'onorevole Verini, segretario regionale umbro del PD, appena qualche settimana fa nel rispondere a un'interrogazione.

magari con sensibilità differenti, hanno fatto presente che all'articolo 59 è ingiusto - e non possono essere ingiusti il Parlamento e il Governo - dire che aiutiamo le attività economiche dei centri storici delle città d'arte a vocazione turistica, ma solo

da tutti i partiti politici. Dovrei fare una classifica, che il tempo non mi consente, dei Comuni danneggiati. Mi limito a citarne uno, da dove il 14 agosto siamo partiti e con i colleghi Borgonzoni e Centinaio abbiamo

quando si hanno a disposizione 25 miliardi di euro e l'intero Parlamento chiede un intervento, è ingiustificabile. *(Applausi)*.

Se infatti non ci fosse stato l'intervento - sottoscritto da tutti i Gruppi, ma presentato a mia prima firma per la Lega - per evitare il blocco della raccolta differenziata e il conferimento in discarica, avremmo avuto tutto fermo dal 29 settembre.

la tabella 5A, invece della tabella 5, mettendo di fatto fuorilegge il conferimento dei rifiuti urbani in discarica. Se, dunque, non avessimo corretto noi questo errore, si sarebbe bloccato tutto. Sarà importante quindi - io dico - che in una Repubblica parlamentare ogni tanto il Governo, oltre che dopo aver commesso un errore come in questo caso, ma anche prima, ascolti un po' più il Parlamento, soprattutto quando tutti i Gruppi sono d'accordo per evitare che i problemi si creino? Potrei andare avanti ancora molto. Faccio solo un breve riferimento a quanto si sarebbe potuto fare e non si è fatto, ma che si potrà fare nel collegato ambientale, dove l'inammissibilità non c'è: sblocchiamo una buona volta la chiusura del ciclo dei rifiuti con l'utilizzo del combustibile solido secondario. Tutti i Gruppi sono d'accordo, tranne uno. Questo è un esempio, ma ce ne sarebbero altri. L'Italia non merita tutto questo, non merita che un singolo Gruppo parlamentare, soprattutto in materia ambientale, blocchi tutti gli altri. Non lo meritano gli italiani di oggi e di domani, visto che il conto dei 25 miliardi lo pagheranno anche

cioè, ad evitare la chiusura del suo salone di acconciatura per signore ereditato dal padre, un pezzo di storia ormai quarantennale in uno dei quartieri storici di Roma? Perché l'attività va, sì, avanti, ma a singhiozzo. Questo maledetto coronavirus, che sta stravolgendo la vita della gente, rischia di mettere in ginocchio anche l'azienda di Fabio e, insieme alla sua, quella di 90.000 altri imprenditori, che, senza aiuti da parte del Governo, rischierebbero di chiudere, causa Covid-19. Per lo più, si tratta di aziende che, con grandi sacrifici, stanno cercando di fare l'impossibile per evitare la chiusura. Ecco che questo decreto-legge rappresenta un ulteriore passo importante per andare incontro a imprenditori come Fabio e fronte alla drammatica situazione nella quale il nostro Paese ancora si trova. Innanzitutto, assegniamo risorse vere, più di 25 miliardi di euro, che portano i fondi complessivamente stanziati dall'Italia dall'inizio della pandemia ad oggi a 100 miliardi, soldi di cui il nostro Paese ha urgentemente bisogno per far fronte agli effetti della crisi innescata dal Covid-19 e finanziare misure che servono a sostenere l'occupazione e garantire quella liquidità che come Italia Viva abbiamo chiesto sin dall'inizio del coronavirus per sostenere chi lavora e chi crea lavoro lavoro e che quindi aiuta la gente, le imprese, i lavoratori e le famiglie ed è in grado di assicurare nel breve termine la tenuta della nostra economia. Con questo provvedimento ripristiniamo il *jobs act*, una misura che avevamo introdotto a suo tempo col Governo Renzi e che ha portato a risultati di grande impatto: un incremento dell'occupazione di oltre 650.000 unità in appena un anno e mezzo ed il calo della disoccupazione giovanile nello stesso periodo di ben sei punti percentuali; il tutto attraverso la decontribuzione delle imprese che assumono in modo stabile e ciò equivale a dire che lo Stato, per un certo periodo, si fa carico del versamento dei contributi previdenziali per i neoassunti che le aziende occupano a tempo indeterminato. Lo Stato, quindi, aiuta le aziende a investire nelle persone, esonerandole dal pagamento degli oneri contributivi: è una misura che ha saputo rilanciare l'economia ed è positivo che la riproponiamo ora, di nuovo, per aiutare le aziende a creare nuovi posti di lavoro stabili e sicuri. una formula vincente anche per il Sud, dove le imprese, con questo decreto, potranno godere di una detassazione del 30 per cento in caso di nuove assunzioni. È una svolta per il Mezzogiorno e un modo per distaccarsi dall'assistenzialismo fine a sé stesso, rilanciando invece le politiche a favore del lavoro e della crescita, per offrire prospettive di futuro ai tanti talenti del Sud Italia che troppo spesso si sono visti costretti a intraprendere la strada dell'emigrazione. Questo decreto-legge ci consente, al contempo, di rafforzare anche le tutele sociali, soprattutto a favore delle famiglie e dei soggetti più vulnerabili, che sono usciti particolarmente provati da questa pandemia. Penso innanzitutto all'estensione temporale del *bonus baby sitter*, voluto dal ministro Bonetti, una misura che aiuta migliaia di genitori alle prese con i problemi causati dal coronavirus a coniugare con maggiore facilità lavoro e vita familiare, consentendo a entrambi i genitori di continuare a lavorare grazie al ricorso a *baby sitter* occasionali, anche durante mesi complicati come questi, legati al rischio di contagio da coronavirus, in cui i bambini possono essere costretti a stare a casa, nell'impossibilità, tra l'altro, di venire accuditi dai nonni. però anche all'introduzione del *bonus* casalinghe, un contributo *una tantum* rivolto alle donne che vogliono qualificarsi e che adesso si occupano dei lavori domestici, oppure della cura dei figli o di familiari malati: una somma attraverso la quale migliaia di donne avranno la possibilità di frequentare un corso di formazione e di conseguire qualifiche lavorative che consentano loro il ritorno o l'ingresso nel mondo del lavoro. Prevedere lo stanziamento di 3 miliardi per la formazione professionale delle donne non occupate è una scelta strategica, perché il rilancio del nostro Paese può passare anche attraverso una maggiore inclusione delle donne nel mondo del lavoro. Il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a convertire prevede, insomma, una serie di misure volte a favorire il rilancio dell'economia, come ad esempio per le attività legate al settore turistico e alla ristorazione, soprattutto quelle situate nei centri storici, spesso piccole e micro imprese che continuano a soffrire fortemente della situazione legata al coronavirus. Grazie all'impegno del ministro Bellanova siamo riusciti, ad esempio, a prevedere l'istituzione di un fondo per la ristorazione, 600 milioni di euro per contributi destinati a ristoranti, pizzerie e trattorie, ma disponibili anche per mense, per agriturismi dotati di attività di ristorazione e imprese che svolgono *catering* continuativo per eventi. Le risorse a fondo perduto dovranno essere spese per acquistare prodotti alimentari tassativamente *made in Italy*: in tal modo, non solo si contribuisce a sostenere le attività di ristorazione che in questi mesi hanno subito perdite ingenti, ma si sostiene anche l'intera filiera agricola del nostro Paese, martoriata dal crollo dei consumi nel settore della ristorazione. Si tratta insomma di un decreto-legge molto ampio, con numerosi ambiti d'intervento, allo scopo di affrontare e alleviare le tante difficoltà in atto. Mi preme sottolineare però in particolare tre ulteriori dettagli, di cui si è arricchito il provvedimento nel corso dell'*iter* parlamentare, grazie anche all'impegno di Italia Viva. Si reintroduce la possibilità per i contribuenti di devolvere il 2 per mille delle proprie tasse, in sede di dichiarazione dei redditi, a favore di un'associazione culturale. Si tratta di uno strumento già sperimentato nel 2016, con il Governo Renzi, che aveva dato prova di grande utilità nell'individuare risorse alternative per il mondo dell'arte, della musica, dell'archeologia, del cinema e del teatro. uno strumento che, a maggior ragione, può risultare strategico adesso, in una fase così difficile in cui proprio il mondo della cultura paga un prezzo altissimo a causa del crollo del turismo e della mobilità. Proprio per aiutare a superare queste difficoltà, ci siamo battuti affinché si riconosca anche un beneficio fiscale alle imprese che operano nell'intero settore dello spettacolo dal vivo, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese effettuate: è un risultato importante, per un settore duramente colpito dalla pandemia. Siamo contenti poi di poter tirare finalmente un sospiro di sollievo: la Casa internazionale delle donne non chiuderà. Dopo mesi di tribolazioni e di ansie, finalmente possiamo rassicurare le tante persone che si sono mobilitate per impedirne la chiusura. Grazie al gioco di squadra con altre forze politiche, è stato possibile infatti approvare un nostro emendamento che, attraverso lo stanziamento di idonee risorse, mette in sicurezza i conti e consente di estinguere il debito pregresso nei confronti di Roma Capitale. In sintesi, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare è una misura a 360 gradi, con aiuti e impulsi: aiuti per chi, come Fabio, si trova in particolare difficoltà in questa fase. *(Applausi).*

È questo un elemento che ci dovrebbe sempre caratterizzare, al di là delle fasi e delle parti politiche che ciascuno di noi ricopre.

contiene innovazioni rispetto all'origine, su cui poi mi soffermerò, ma soprattutto avviene in un contesto nel quale c'è la consapevolezza di tutti di aver lavorato anche con le opposizioni per provare a verificare su alcuni contenuti lo spazio per creare una scelta comune.

che si è protratta, ma che si protrae oggettivamente sul terreno del lavoro, delle imprese, delle famiglie e dei consumi, che ha bisogno di questi interventi. Credo che Credo che per ciascuno di noi, ma soprattutto per chi ci ascolta e per il popolo italiano, dalle imprese alle famiglie, ai lavoratori e al mondo in generale, basti andare a vedere l'insieme degli interventi perché già si configuri il fatto che lo Stato e questo Parlamento, votando

io - della globalizzazione. A volte non ci rendiamo nemmeno conto che c'è un disallineamento fortissimo per l'Italia, che è un Paese

sicurezza sul lavoro, coniugandolo con occupazione e crescita. Qui unifichiamo questi temi ed è fondamentale la tutela del posto di lavoro in sicurezza. Guardate quanto dibattito negli anni precedenti abbiamo fatto per distinguere più crescita,

ha introdotto. Sono esattamente per presentarlo così, perché è un'ulteriore aggancio nelle fasi successive: quello di sapere che puntiamo alla tutela dei diritti delle persone dentro i luoghi di lavoro, perché sono parte qualificante degli elementi di competitività dell'economia reale in tutto il sistema produttivo. In questo c'è anche un'innovazione - ripeto - di cultura politica, industriale e del lavoro, che considero importante.

mi auguro - anche alla Camera. A tale proposito, signora Presidente, vorrei fare un grande augurio ai deputati e alle deputate che purtroppo sono stati contagiati dal Covid-19 perché, anche da questo punto di vista, non si fermino mai i lavori parlamentari, né al Senato, né alla Camera. Credo che ci sarà una discussione nelle Aule del Senato e della Camera che immediatamente dovrà intrecciare le priorità e i contenuti che vogliamo portare dentro le strategie di attuazione del *recovery fund*, quindi nel famoso *recovery plan*.

fare investimenti a sostegno di luoghi come la Casa internazionale delle donne, che operano da anni per sostenere e contrastare la violenza sulle donne, non è una marchetta, termine proprio

voglio ricordare che le cifre delle quali ho sentito parlare in Aula non sono assolutamente quelle reali previste dal provvedimento.

Lo diciamo perché la cifra non è 3 miliardi per le casalinghe e i casalinghi. Se chiamiamo Pierino

ha questo male e se lo trascina. Vorrei dare invece una cornice e un corredo, se me lo consentite, di riferimenti valoriali antagonisti rispetto a quelli che ho visto emergere nel provvedimento,

delle teorie marxiste. Abbiamo visto quanto accaduto in altri Paesi e credo di poter dire, senza tema di smentita alcuna, che, se Carlo Marx, sostenitore di certe teorie, tornasse qua, direbbe immediatamente: proletari di tutto il mondo, non unitevi, ma perdonatemi, perché le teorie che sono state

mercato, le imprese, l'intrapresa, il rischio e coloro che hanno il coraggio di affrontare il mercato in una situazione di estrema difficoltà come quella che si sta attraversando. Questo provvedimento complica e non semplifica. Abbiamo una burocrazia soffocante per gli imprenditori. Lo voglio annunciare, purtroppo, anche ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti e a coloro che sono nel menù delle necessità di questo Governo. Governo. Ci troviamo di fronte a un'emergenza particolare, in cui gli assistiti sono molti di più rispetto agli assistenti, cioè coloro che dovrebbero produrre reddito. Questa situazione è davvero di enorme difficoltà. Di fronte a uno Stato di polizia tributaria, come quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti,

della libertà d'impresa. Avremmo dovuto aiutare gli imprenditori, non fare politiche assistenzialiste. Voglio ricordare l'intervista che Draghi ha rilasciato al «Financial Times» nel mese di marzo di quest'anno, mi pare. Ha evidenziato la necessità

si tratta di redistribuzione del reddito; avremmo impiegato meglio le nostre risorse se avessimo aiutato le imprese e soprattutto avessimo abbassato le tasse, se si fosse andati verso la *flat tax*, se avessimo

velocità di circolazione della moneta e, se questa viene bloccata, ovviamente si inceppa anche il meccanismo di crescita. Penso allora all'abbassamento delle tasse,

l'edilizia: da lì si dovrebbe ripartire, non dai *bonus* vacanza o da *bonus* dati a pioggia che poi non sortiscono alcun

detto che sulla riviera romagnola sono in vendita 300 hotel, imprese importanti che erano il tessuto connettivo portante della nostra Nazione, pronte a prendere il volo verso altre direzioni. Avviandomi sento parlare di rimbalzo, mi viene un po' il sorriso sulle labbra e mi chiedo da dove rimbalziamo. Dopo tre mesi di chiusura, è chiaro che un rimbalzo c'è stato, ma dipende sempre da dove si parte.

l'ennesimo decreto-legge che non porterà nulla di concreto ai cittadini e che si porterà dietro altri decreti attuativi che non arriveranno mai e, se arriveranno, magari sarà troppo tardi. Sono i dati a confermare che le misure adottate sino ad oggi sono state inefficaci per contrastare la crisi economica dovuta al Covid: il calo del PIL dell'8 per cento ci fa capire che non hanno sostenuto le aziende e la loro produzione. L'Istat stesso ha evidenziato che, mentre il reddito degli italiani è diminuito, le tasse sono aumentate e le bollette sono schizzate alle stelle. Le toppe che ad oggi avete cercato di mettere, in molti casi, si sono rivelate peggiori dei buchi stessi. Provate ad andare a parlare con la gente comune, con chi ha una partita IVA o con chi la mattina alza una saracinesca, e chiedete loro che cos'è arrivato dal Governo per far fronte all'emergenza. Vi risponderanno che sono Hanno pagato tutti le tasse, magari hanno anticipato la cassa integrazione ai dipendenti; chi aveva qualche risparmio - i sacrifici di una vita - lo ha dilapidato. Qualcuno non ha riaperto l'attività; qualcuno ha riaperto fiducioso, ma a settembre ha chiuso i battenti, magari dopo quarant'anni di duro lavoro e con la difficoltà di potersi ricollocare.

Abbiamo danni ingenti, stimati intorno ai 30 milioni, e vittime; quest'emergenza va a sommarsi alle altre, dal crollo del ponte Morandi

se le emergenze gestite dalla Regione hanno avuto soluzioni rapide, quelle del Governo centrale tardano ad arrivare e molto spesso peggiorano situazioni già critiche. Il vostro grado di efficienza nel trovare rapide soluzioni a ciò che accade è a un chilometro da casa mia. Parlo del ponte di Albiano, crollato l'8 aprile scorso, dov'è evidente la gara di inerzia tra il Governo, la Regione e il Comune. Ad oggi non si è stati in grado di rimuovere un sasso dall'alveo del fiume; non vi è neanche la minima idea di un progetto per la ricostruzione, ma nel frattempo sono stati nominati tre commissari. Abbiamo danni all'economia locale, disagi negli spostamenti sia per gli studenti sia per chi si deve recare al lavoro, oltre all'angoscia dei cittadini che vivono ai lati del fiume per possibili allagamenti che potrebbero avvenire a causa dell'effetto diga per le macerie in alveo; ma, anziché fare un *mea culpa* per ciò che evidentemente non siete stati in grado di fare in ogni ambito (dalle infrastrutture alla gestione dell'emergenza Covid, al

emergenze e, anziché ricevere critiche, dovrebbero avere il supporto da parte del Governo. al decreto-legge agosto, oggetto di questa discussione, ho presentato come prima firmataria un emendamento all'articolo 11 (quello contenente misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'arsenale militare

Poiché articolo 11 ed emendamento sono identici nei contenuti, vorrei capire come si può dichiarare inammissibile un emendamento pressoché uguale all'articolo a cui fa riferimento. È evidente l'arroganza di questa maggioranza che, senza alcuno scrupolo, boccia gli emendamenti presentati dall'opposizione esclusivamente per scelta politica e non per contenuto o per mancanza di fondi. Oltre a privare le due Camere di dignità, siamo arrivati a rendere inutile anche il lavoro delle Commissioni. La richiesta di nuove assunzioni in tutti gli arsenali militari arriva dal Capo di stato maggiore della Marina, che ha evidenziato come il numero ridotto di personale presente, abbinato ai prossimi pensionamenti e al numero di anni necessari alla formazione di nuove maestranze, porterà a breve al collasso di tutto il sistema, con il rischio concreto di dover esternalizzare quanto oggi invece riusciamo a realizzare con le nostre professionalità.

Tutti avevano le medesime criticità legate all'occupazione, non solamente quello di Taranto. Tutti hanno la stessa dignità.

Inutile è stato il lavoro della Commissione, perché, come abbiamo visto, l'emendamento è stato bocciato. In pratica, viene considerato solamente l'arsenale di Taranto.

conseguenza delle trattative che ci sono state per l'assegnazione delle Presidenze delle Commissioni. Questo nulla ha a che vedere con il bene della Nazione. Mi stupisco dei colleghi liguri, che hanno accettato silenziosamente questo affronto alla nostra Regione, che fanno parte della Commissione difesa e che hanno privato il loro territorio di risorse per questioni puramente di convenienza

È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà. il decreto-legge che stiamo per approvare riversa altri 25 miliardi di euro nel sistema Paese, facendo arrivare a 100 miliardi la cifra complessiva stanziata per far fronte alla crisi economica. Gli interventi riguardano molti settori, che spaziano dal lavoro alla coesione territoriale, alla salute, alla scuola, alle Regioni e alle misure economiche e fiscali per sostenere l'economia. In questo, come negli altri decreti approvati sinora, emerge prepotentemente che lo Stato c'è e sostiene i suoi cittadini. *(Applausi)*. Gli interventi a favore dei lavoratori di Air Italy, concessi nell'articolato, illustrano bene i paradossi a cui è andato incontro in passato il settore aereo. Questa compagnia privata, nata nel 2018, non è mai decollata e ha chiuso l'attività nel febbraio 2020, per cause indipendenti dall'epidemia: semplicemente i ricavi non compensavano gli investimenti, malgrado di interventi pubblici regionali e, in definitiva, statali a sostegno di una società privata. Il privato ha abbandonato lo scalo, lasciando a terra 1.500 dipendenti. Immediato è il confronto con l'Alitalia, che molti vogliono privatizzare da tempo. Tutte le compagnie aeree hanno subito un pesante contraccolpo ed è evidente che, in questo momento, nessuna possa farcela da sola. Molti si lamentano che abbiamo speso miliardi di euro per sostenere l'Alitalia, ma dimenticano che, accanto all'industria, il turismo è una delle principali fonti di introito del Paese e una compagnia di bandiera, che alimenti il settore, è indispensabile. Il bilancio sembra in perdita, ma chi ne usufruisce sono le migliaia di esercizi commerciali sparsi nel territorio. Un mero calcolo, basato sulle spese e sulle perdite di una compagnia aerea, non può e non deve essere l'unico elemento di valutazione. Nel caso di Air Italy, un buon Governo non lascia sul lastrico 1.500 famiglie. Chi è fautore del libero mercato potrebbe sostenere che, per una questione di equa concorrenza, anche i privati debbano usufruire delle stesse agevolazioni delle compagnie di Stato. Si dimentica tuttavia che spesso accade il contrario, cioè che le compagnie private, le *low cost*, ricevono ingenti agevolazioni regionali, che in definitiva sono statali, solo pubblicizzate con meno clamore, e spesso si applicano alle compagnie di bandiera tariffe superiori a quelle delle *low cost*, perché per le compagnie statali paga lo Stato. Anche i dipendenti di altri settori del trasporto, spesso in mano a privati, come quello marittimo, hanno ricevuto un aiuto importante e un intervento significativo è rivolto anche alle compagnie che si occupano di trasporto pubblico locale e ferroviario, che ancora stenta a riprendersi, a causa dei vincoli stringenti imposti dal distanziamento fisico. Ricordo che, durante la fase acuta dell'emergenza, sia Alitalia sia Ferrovie dello Stato hanno garantito i trasporti essenziali per riportare a casa i nostri concittadini e garantire la consegna delle attrezzature mediche, che hanno salvato tante vite umane. È ovvio che lo Stato debba in tutti i modi tutelarsi e prevedere liquidità a fronte dell'effettiva diminuzione di fatturato di un'impresa e infatti, nel capo I, il contributo per la cassa integrazione è fornito in funzione delle percentuali di riduzione di fatturato. È altrettanto ovvio che siano necessari controlli. Le opposizioni si lamentano del reddito di cittadinanza, definendolo una misura assistenziale, ma quando è scoppiata la pandemia si era tutti concordi nel chiedere l'immediatezza degli aiuti, invocando controlli solo *a posteriori*. Il reddito di cittadinanza ha svolto una preziosa funzione di ammortizzatore sociale, per milioni di nullatenenti, evitando rivolte di piazza, alimentate dalla disperazione Pensate che tutti i liberi professionisti o tutte le imprese a cui è stato dato un contributo abbiano subito perdite reali? L'INPS e il tanto vituperato presidente Tridico, che ringrazio pubblicamente per l'abnegazione e la competenza dimostrate hanno avviato procedure di controllo, individuando migliaia di tentativi di frode. Gli italiani dovrebbero sapere che la cassa erogata impropriamente per il Covid sembra ammontare a circa 2,7 miliardi mentre le piccole truffe del reddito cittadinanza sono costate 4,5 milioni di euro: non c'è paragone! L'articolo 46 stanzia oltre 2,65 miliardi di euro a favore dei Comuni per opere pubbliche e la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Mai come in questi giorni, dopo l'emergenza maltempo che ha colpito il Nord-Ovest, ci rendiamo conto di quanto queste misure siano essenziali. Riguardo la proposta di legge menzionata prima dal collega Bergesio, si sottolinea come gli interventi gli interventi non possano essere dati ai singoli Comuni. Il fiume è un ecosistema delicato, che necessita di interventi oculati lungo tutto il tratto.

perché non abbiamo fatto leggi lo scorso anno. Io chiedo perché chi ora è all'opposizione non l'abbia fatto nei decenni precedenti. Per decenni i Comuni sono stati trattati come nemici da abbattere, dato che il Comune è la più antica forma di partecipazione democratica: nei Comuni i rappresentanti dei cittadini continuano a essere eletti direttamente dalla cittadinanza, cosa che il MoVimento 5 Stelle continua a ritenere indispensabile per una nuova legge elettorale. Lo strangolamento dei Comuni, realizzato tramite la progressiva decurtazione degli stanziamenti, è stato un atto deliberato dei vari Governi che ci hanno preceduto. Ogni Gruppo politico in quest'Assemblea faccia un *mea culpa*, perché sono pochi quelli che non hanno sostenuto questa politica. È stato solo con i Governi Conte che un po' di ossigeno è fluito nuovamente verso i Comuni e gli enti locali e sono state stanziate risorse per la messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici. Con l'articolo 48 anche le Città metropolitane e le Province sono destinatarie di un finanziamento di 1,125 milioni di euro per l'efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici. Con l'articolo 49 si prevedono finanziamenti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli non sicuri. Le strade sono state finanziate, dopo decenni di mancata manutenzione che hanno sicuramente pesato sulla salute dei cittadini. Con l'articolo 50 vengono, invece, semplificate le procedure per gli interventi di rigenerazione urbana, un tema estremamente caro al MoVimento, che da sempre sostiene la necessità di diminuire il consumo di suolo e di avviare la riqualificazione delle aree abbandonate, che in molte città diventano periferie degradate. Viene inoltre istituito un fondo per l'adozione di specifiche strategie per l'abbattimento dell'inquinamento nella Pianura padana, dato che il cancro ai polmoni interessa un uomo su nove e una donna su trentasette. Il tumore ai polmoni uccide 80 italiani al giorno; l'incidenza è, però, enormemente superiore nella Pianura padana, in quanto la forte industrializzazione è spesso carente del rispetto delle norme in materia di emissioni. Troppo spesso l'industria che inquina viene perdonata perché crea lavoro; spesso i cittadini non se ne rendono conto, pur essendo coinvolti. Doveva arrivare il MoVimento 5 Stelle per intervenire pesantemente su questa situazione. Con l'articolo 51 sono previsti investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, anche per l'abbattimento di barriere elettroniche. Arriviamo, poi, all'articolo 57, che si occupa nuovamente delle aree terremotate. Vari articoli si occupano di mobilità dolce, perché con questo Governo stiamo spingendo l'acceleratore verso una nuova Italia, una nuova Europa, con un'economia basata sulle energie rinnovabili. Cerchiamo di ridurre l'impatto delle emissioni di CO2 nell'atmosfera e di fermare il cambiamento climatico; è anche questo un cambiamento epocale. Avevamo annunciato delle rivoluzioni e le stiamo attuando. Per bloccare in maniera consistente il cambiamento climatico è, però, necessario un nuovo modello di sviluppo, che dia priorità all'economia circolare, che abbatta i consumi superflui e gli sprechi alimentari e per ridurre le disparità economiche e sociali, che creano Regioni a velocità di sviluppo differenziato anche all'interno del Paese. Credo che la politica sia una cosa seria e, al di là delle facili demagogie, questo Governo ha emanato una serie di provvedimenti che tendono veramente a semplificare le procedure burocratiche e amministrative e contemporaneamente mettono mettono in circolo cifre ingenti per l'ammodernamento del Paese e il sostegno di imprese e cittadini, processo che non cesserà fino a quando al Governo ci sarà il MoVimento 5 Stelle. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, sono molto d'accordo con l'impostazione che è stata esposta dai relatori e nei molti interventi che mi hanno preceduto e quindi la voglio riprendere.

giustamente interviene sui lavoratori fragili e su tutte quelle fragilità su cui è necessario intervenire per - noi diciamo (e questo è un punto di impostazione) - parlare seriamente di ripartenza. Non è semplicemente un dovere etico e morale o una concezione delle nostre comunità; è un obiettivo che nasce dal

alla presa d'atto del fallimento di un modello di sviluppo basato sull'austerità e sull'individualismo e della necessità della riconversione su una serie di settori che mettano al centro la coesione sociale, il *welfare,* la ormai sufficientemente ricordata transizione ecologica, la ricerca e - ultimo, ma non ultimo - il ruolo delle donne nella società.

alle politiche pubbliche che, di nuovo, è un grande elemento di innovazione, con un'idea del ruolo in Europa e di quello che si può ottenere dall'Europa che è diversa dall'idea del tiro alla fune in Europa per ottenere

dai toni anche aspri; sappiamo che è una battaglia ancora non completamente vinta. Quindi, no al tiro alla fune e sì all'opportunità di progettare un nuovo mondo che veda

dell'idea per cui la transizione ecologica fa parte di questo concetto largo di cura ed è oggi più che mai assolutamente collegata e inscindibilmente connotata dall'idea di una nuova politica industriale e di una tecnologia molto avanzata. In sostanza, noi oggi non possiamo parlare di questi argomenti se non li sposiamo con la tecnologia. la tecnologia. Dare questa direzione alla tecnologia è per un verso una scelta e per un altro verso è una sfida. È stato anche ricordato, non solo oggi in quest'Aula poiché è un argomento di dibattito pubblico con toni dialettici accesi, il rapporto e il ruolo dell'opposizione rispetto alle scelte di governo

avremo un'occasione molto importante: tra pochissimi giorni c'è la discussione sulle linee del *recovery fund*. Facciamo allora in modo che sia un'occasione per confrontarci davvero su una visione

Ma è altrettanto evidente che di politica fiscale si deve parlare in un quadro generale strategico e di rimodulazione del prelievo fiscale, con delle scelte che usino la leva fiscale. Signor

- permettetemi - rozzo pensare che tutto questo non abbia a che vedere con lo sviluppo della nostra comunità e della nostra società. Se mai, noi pensiamo che questo sia solo un piccolissimo passo rispetto a un quadro più generale che non riguarda solo questa specifica Casa internazionale delle donne, che è a Roma ma che ha un valore nazionale, tant'è vero che abbiamo presentato alcune proposte di legge,

bisogno per tutta la collettività, e non ovviamente solo a tutela delle donne. Signor Presidente, membri del Governo, a quota 100 miliardi di indebitamento netto. Questo è esattamente quanto Forza Italia e i responsabili economici avevano chiesto all'inizio di questa crisi come misura rispetto alla quale ci saremmo confrontati per mettere in campo Non è stato possibile. Avete condotto una politica fatta di una successione di decreti - siete arrivati adesso a 100 miliardi di indebitamento perché evidentemente la visione che avevate e che avete tuttora non vi ha consentito di prevedere queste cose per tempo, tant'è che oggi praticamente dovete comunque intervenire con misure di sostegno al reddito dentro i 25 miliardi. La battuta sarebbe scontata: non c'è solo il reddito di Tridico in discussione; ci sono situazioni ben più gravi e ben più importanti. La cassa integrazione straordinaria ancora non è arrivata in modo omogeneo nel Paese. È Paese. È stata poi introdotta una misura assolutamente nuova, ma solo per alcune Regioni italiane: la fiscalità di vantaggio solo per il Sud, mentre il resto del Paese è estraneo a questa vicenda. Il costo del lavoro e la nostra capacità di essere competitivi in Europa e nel mondo passano in secondo

con due Paesi dell'Unione europea, dove la *flat tax* esiste da tempo e dove la fiscalità di vantaggio è una necessità per contenere la delocalizzazione.

Il problema della casa è centrale. Abbiamo chiesto e chiediamo con forza l'introduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali; lo avete annunciato, ci sono stati più interventi all'interno della maggioranza, che sono dissipati, non si sono visti. Abbiamo proposto un emendamento che veniva incontro a questa esigenza, dicendo ai proprietari di ridurre il canone a fronte del vantaggio di una riduzione della cedolare, ma non lo avete accolto.

delle procedure di sfratto, che nulla hanno a che fare con la vicenda della pandemia, perché sono maturate precedentemente. rispetto a questo quanto meno avreste dovuto prevedere un fondo di indennizzo per quei proprietari che integrano la pensione o che ricevono il reddito semplicemente dalla locazione e non possono riceverlo perché sono bloccati da un anno e più nelle

Fortunatamente so che in Commissione bilancio si è prevista la possibilità di estendere fino fino a dicembre 2020 la cessione del credito per le locazioni degli alberghi: va benissimo, ma questa doveva essere una misura concepita per tutte invece non lo avete fatto. Costava 500 milioni di euro: all'interno di 25 miliardi non siete riusciti a concepire questa misura, non siete riusciti a concepire una misura che rimetta in moto il mercato immobiliare, che risolva un problema annoso. Bisognava pensare a rinviare - e il Parlamento avrebbe dovuto farlo - il pagamento della seconda rata dell'IMU: era necessario e si poteva portare a marzo L'IMU continua a dare allo Stato un gettito di 22 miliardi. Dal 2012, per effetto di una misura voluta dal professor Monti, abbiamo aumentato in modo indiscriminato i coefficienti catastali. Il risultato è che sulla casa, sull'immobiliare, grava una tassazione senza precedenti, asfissiante, che è di fatto un blocco alla nostra economia. Su le tasse sulla casa, giù i valori immobiliari: questo è stato l'impoverimento degli italiani, rispetto al quale, con le misure opportune che vi abbiamo suggerito, avreste potuto dare ossigeno ad un settore

e da altre colleghe che mi hanno preceduta, soprattutto in tema di *welfare*, di politiche a sostegno delle famiglie e, di conseguenza, a sostegno delle donne anche dal punto di vista occupazionale

emancipazione e dal loro ingresso nel mondo del lavoro, perché sono quelle che sicuramente hanno sofferto di più, in questo periodo lunghissimo di *lockdown* e di pandemia, che purtroppo non è ancora finito. quindi, delle misure importanti; non si può dire che non ci sia qualcosa di positivo in questo provvedimento. Ci sono delle azioni concrete, ci sono delle misure economiche a sostegno proprio di quei settori strategici

considerato un aspetto marginale. Sappiamo, invece, come sono aumentati, purtroppo, i casi di violenza sia sulle donne che sui minori proprio all'interno delle famiglie, anche a causa di questo permanere dei contagi da Covid. quindi, sono misure che vanno ad aiutare e a sostenere anche questo aspetto, che per noi rimane fondamentale. Certo non risolve i problemi, perché sappiamo che servono misure strutturali, ma infatti nei prossimi giorni parleremo di *recovery fund*

soprattutto se ci sarà la proroga dello stato di emergenza. È necessario fare un dibattito - lo abbiamo detto in questi giorni - all'interno del Parlamento, nelle Aule parlamentari, prendere tutte quelle risorse e e spenderle bene sia per quanto concerne il *recovery fund*, sia per quanto riguarda il MES. L'altro aspetto che vorrei sottolineare rapidamente riguarda due due emendamenti di Italia Viva che sono stati approvati in questo decreto-legge, di cui parlava bene prima la senatrice Garavini e che interessano la mia Commissione,

In questo senso, i due emendamenti che sono stati approvati cominciano a rimettere al centro anche il patrimonio culturale di cui è ricco questo Paese. E quando parliamo di cultura parliamo anche di rilancio economico perché stiamo parlando di un patrimonio straordinario ed unico che ha l'Italia nel mondo. In questo senso sono stati approvati due emendamenti che considero molto importanti. *tax credit*, che significa appunto riconoscere un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese effettuate dalle imprese che svolgono attività inerenti all'intero settore dello spettacolo dal vivo. Questa proposta mira proprio a dare un sostegno concreto a questo settore che è stato duramente colpito dalla pandemia. Per quanto riguarda il 2 per mille, è una norma che era stata varata nella legge di bilancio del 2016 dal governo Renzi e che oggi, grazie all'emendamento di Italia Viva, è stata approvata all'interno di questo provvedimento. Ciò significa un'occasione davvero unica per destinare un contributo

il tema dello sport e della capienza nei palazzetti e negli stadi, che non è un tema secondario, perché lo sport appartiene all'economia e all'imprenditoria di questo Paese. Vorrei concludere dicendo che iniziamo a parlare di argomenti e di settori che hanno sofferto troppo e a cui con questo provvedimento si cominciano a dare delle risposte concrete. Ci auguriamo che nei prossimi giorni si possa entrare nel pieno dell'azione concreta di rilancio di questo Paese con la discussione sul *recovery fund* e poi il tanto auspicato per Italia viva MES.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, gli ultimi dati che riguardano il numero di rapporti di lavoro rilevano la gravità della situazione in Italia. Essi sono indicativi anche delle politiche economiche e ci sono troppe norme adottate finora dal Governo che irrigidiscono il mercato del lavoro: dal decreto cosiddetto dignità al reddito cittadinanza, che manca l'obiettivo di portare a lavoro chi lo percepisce. decreto agosto oggi purtroppo procede nella medesima direzione, cioè l'assistenzialismo, ma mancano le cosiddette politiche attive. Più di un milione di posti di lavoro persi, una cifra che senza una chiara inversione di tendenza, quando finirà il blocco dei licenziamenti, potrebbe anche aumentare. Si stanziano ulteriori risorse (mi dispiace che manchi il ministro Catalfo, con il quale abbiamo più volte colloquiato circa il reddito di cittadinanza):

Lo sgravio del 30 per cento sui contributi pensionistici per le aree svantaggiate del Mezzogiorno per il periodo ottobre-dicembre 2020 è una misura che in realtà lascia forti perplessità, perché si tratta di politiche meramente assistenzialistiche, che peraltro attendono il via libera dalla Commissione europea. Circa un miliardo di costi per sostenere sgravi contributivi che proseguono nell'alveo di politiche disancorate da un disegno di crescita strutturale del Mezzogiorno, perché gli sgravi contributivi erano totali e non limitati al 30 per cento nel Mezzogiorno e furono vigenti fino al 1994, per circa venticinque anni, e furono allora bocciati proprio dall'Unione europea che promosse una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. venticinque anni però non si registrarono incrementi occupazionali; quindi non è una misura nuova e non è nemmeno di portata storica, come si è detto. Nulla per tentare di colmare il cronico divario infrastrutturale del Mezzogiorno, delle isole e ancora più della Sardegna, che sconta, oltre alla discontinuità territoriale, anche l'extra-costo dell'energia. Vengono prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza, ma va purtroppo rammentato che la gestione della cassa integrazione ha lasciato per mesi centinaia di migliaia di lavoratori senza stipendio e senza assegni anche per via delle complesse procedure burocratiche previste. Mancano all'appello più di 100.000 lavoratori. Va altresì ricordato che il 70 per cento degli assegni di cassa integrazione pagati devono ancora essere rimborsati ai datore di lavoro che li hanno anticipati ai lavoratori. Il decreto contiene l'ulteriore misura per le aziende che ora assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta, che prevede l'esclusione del versamento dei contributi previdenziali per un massimo di sei mesi dall'assunzione fino al 31 dicembre. Insomma, un'altra misura temporanea e non risolutiva. Come si può, in questo momento di crisi senza precedenti, pensare che le aziende debbano assumere a tempo indeterminato? La prima preoccupazione che dovrebbe avere il Governo è quella di togliere i lavoratori dall'assistenzialismo e farli tornare alla dignità di avere un lavoro e un salario. Rimane preclusa la via delle procedure di licenziamento individuali, così come sono sospese le procedure di licenziamento collettivo. Vale ricordare che sono circa 400.000 i licenziamenti tutt'ora bloccati e bisogna rilevare che il posto di lavoro non si può mantenere per legge, ma prevedendo misure concrete per fare in modo che la ripresa dell'attività economica produca il reintegro dei lavoratori, ma soprattutto consentire che l'attività economica continui in sicurezza con le protezioni e precauzioni dovute, scongiurando nuove chiusure. Diceva il mio collega Aimi che non possiamo permetterci un secondo *lockdown*. È assolutamente vero. Invece è presente anche la disposizione per cui i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite complessivo di ventiquattro mesi e per una sola volta. Noi ci siamo espressi sempre contro la limitazione dei contratti a tempo determinato e l'eliminazione dei *voucher*, sin dal cosiddetto decreto dignità. Il tempo e la pratica applicazione di quelle disposizioni, soprattutto in questo periodo di crisi, ci hanno dato ragione. Noi chiediamo una maggiore liberalizzazione del mercato del lavoro, un ruolo sempre maggiore della formazione continua per far entrare o rientrare i lavoratori nei ruoli per i quali sono formati. Le nostre posizioni sono avvalorate dai dati di Unioncamere-ANPAL che registrano la difficoltà di reperimento di figure professionali adeguate con percentuali che vanno dal 20 per cento per le figure meno qualificate al 40 per cento per quelle in possesso di maggiore formazione. Noi sosteniamo con profonda convinzione il ruolo della formazione continua che deve contribuire a ridisegnare completamente le dinamiche del mercato del lavoro. Si è investito troppo poco in formazione per la quale bisogna coinvolgere il mondo dell'impresa. Rileviamo che per

Il reddito di cittadinanza ha fallito proprio nello scopo di creare posti di lavoro attraverso il *matching* tra domanda e offerta nei centri per l'impiego, tant'è che solo uno su sei di quelli pronti a lavorare ha sottoscritto un rapporto di lavoro. Mentre riteniamo che comunque debbano rimanere misure mirate di contrasto alla povertà. Insomma questo è un decreto con molte risorse per i temi del lavoro, ma con effetti che purtroppo saranno limitati nel tempo e che mancano l'opportunità di introdurre misure strutturali per rendere più dinamico il mercato del lavoro, mercato che passa sicuramente attraverso una crescita dell'economia trainata dalla crescita delle infrastrutture del Paese per il quale i decreti economici del Governo, in oltre sei mesi, non hanno previsto nulla. Noi continuiamo a pensare che le politiche assistenziali siano utili a ridurre il disagio sociale e la povertà mentre è l'impresa l'unica in grado di creare posti di lavoro in cui il ruolo della regolazione e della contrattazione deve avere solo lo scopo di renderlo più dinamico. A questo proposito e a proposito del divario dell'infrastrutturazione, Presidente, in conclusione voglio ricordare di aver presentato alla Commissione un emendamento per quel che concerne la Sardegna. per il Mezzogiorno ma per la Sardegna in particolare la quale sconta ancora l'assenza del gas metano che potrebbe ridurre il costo dell'energia

onorevoli colleghi, il provvedimento completa la serie che va a comporre i fatidici 100 miliardi di indebitamento che stiamo collocando sul mercato a suon di buoni del tesoro. Attenzione! Parlando con molte persone, complice la pessima informazione, ho compreso che molti credono che questi soldi arrivino già dall'Europa, ma il percorso dei fantastiliardi dell'Europa non è che appena cominciato ed è difficile a oggi prevedere quando e se arriveranno i primi soldi. Per ora

peseranno gravemente sulle generazioni future e per questo, a maggior ragione, andavano spesi con cura particolare e, in una prima fase, in emergenza, ma poi con una seconda fase di visione organica del futuro. Ebbene, ciò che ho denunciato nel mio intervento sul decreto rilancio continuo a denunciarlo qui in questo decreto agosto: non c'è visione. Faccio alcuni esempi: l'articolo 21 prevede il fondo per la formazione personale delle casalinghe. Questa vi sembra una misura di urgenza e rilancio?

L'articolo 43 risolve un contenzioso regionale, nello specifico con la Regione Campania. Vi rendete conto? Con una legge dello Stato si risolve un contenzioso regionale. Si potrebbe poi continuare. Già nell'articolato si trovano misure particolaristiche che nulla hanno a che fare con la ripresa. Veniamo ora alla lunga fase emendativa in cui l'opposizione ha mantenuto un comportamento responsabile e costruttivo. A tal riguardo, ringrazio i due relatori, i colleghi Errani e Manca, ai quali riconosco gli sforzi di mediazione tra Governo e opposizioni, tra maggioranza e minoranza, però adesso bisogna guardarsi negli occhi e dirsela tutta: non è questo il modo di procedere. C'era stata assicurata la trattazione di alcuni argomenti importanti con il recepimento di nostri emendamenti in pacchetti condivisi. Per l'analisi di questi pacchetti ci sarebbe stato riconosciuto un tempo congruo per poterli esaminare e, invece, a parte quattro pacchetti arrivati la sera prima della fatidica nottata, tutto è arrivato a inizio seduta, se non durante la seduta nelle ore notturne.

Un detto suggerito da un amico - è un detto di saggezza popolare - recita: il lavoro fatto di notte si vede di giorno. Non è una bella cosa. Infatti, il lavoro è pasticciato, confusionario e gestito con grande difficoltà dagli uffici, costretti a uno sforzo senza senso. Rivolgo un ringraziamento particolare anche a loro. Infatti, nel resoconto leggo che: «Gli emendamenti segnalati non espressamente posti in votazione, né espressamente ritirati o trasformati in ordini del giorno, sono stati

Quegli emendamenti che erano segnalati sono stati valutati dal Governo e dalla maggioranza e sono stati respinti politicamente.

è stato stilato un elenco indicativo e non esaustivo dei Comuni in stato di emergenza per eventi calamitosi. Ebbene, il Piemonte (con altre zone d'Italia) è stato dimenticato: si tratta, cioè, di un errore dell'Agenzia delle entrate.

Non è previsto nulla per i piccoli, nessuna visione d'insieme sulle strutture ricettive, che non sono soltanto grandi alberghi ma anche agriturismi *bed and breakfast*, campeggi, villaggi. Con l'emendamento 99.3 (testo 2) volevamo proporre la sospensione dell'invio di tutte le cartelle esattoriali, la cui partenza - come sapete - è prevista per metà ottobre; non è una pace fiscale ma si voleva bloccare questa partenza. Gli italiani hanno già tanti problemi, lasciamoli vivere, non tartassiamoli con cartelle da cui sovente ci si deve difendere. Anche questo emendamento è stato bocciato, quindi le cartelle partiranno. ad alcune proposte abbiamo trasformato i nostri emendamenti in ordini del giorno, nella speranza che qualcosa venga recepito nella legge di bilancio, come ad esempio la proroga del *bonus* facciate, che non è coerente con la scadenza del *bonus* al 110 un po' di logica: non abbellisco prima la facciata e poi la distruggo per realizzare il cappotto; nel mondo reale funziona esattamente al contrario.

o volete soltanto riempirvi la bocca di rimbalzi che non ci saranno mai (queste sono le parole del ministro Gualtieri)? l'economia non si riavvia con l'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e neanche dando 900.000 euro per la Casa internazionale per sanare un debito con Roma Capitale. È ora di smetterla di fare politica per accontentare questo o quel minimo interesse. Siamo in emergenza economica; cari colleghi, bisogna mettersi in testa che bisogna fare politica per l'Italia e per gli italiani.

- o meglio, il vostro - Presidente del Consiglio è venuto anche in Umbria, nella terra di Francesco, anche lui ha esordito con la sua "enciclica". Non so se lo abbiate ascoltato; ha trattato temi altamente esistenziali a discapito dei problemi di tutti i giorni della gente: «Riscopriamo il valore dell'essenziale, di ciò che è invisibile agli occhi ma decisivo per l'esistenza Questa pandemia ci ha reso coscienti del valore della relazione (...) Abbiamo compreso di essere fratelli tutti (...) Stiamo elaborando un piano nazionale per un Paese rigenerato». Una bella sberla in faccia ai problemi veri degli italiani, ai problemi che tutti i giorni gli italiani incontrano, dai cassintegrati ai commercianti agli operatori delle mille attività economiche che stanno in ginocchio. dei terremotati dei crateri dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, dell'Abruzzo, ai quali destinate in questo provvedimento 15 milioni Un problema che ci trasciniamo da anni ormai; una ricostruzione che non solo non è partita ma non è neanche all'orizzonte, non è neanche anticipata; ancora ci sono le macerie.

Covid abbiamo accumulato una serie enorme di ritardi gravissimi, che comporteranno danni dal punto di vista terapeutico - ormai questo è stato evidenziato da tanti della comunità scientifica - che ci trascineremo

perché non è pensabile che quello che non si è fatto in anni, in una situazione ulteriormente aggravata dal Covid, venga smaltito in tre mesi. Non esiste, è una cosa senza senso, è una cosa fatta a rovescio.

dice che la tabella B differisce da quella risultante dalle somme dell'allegato A, per la scelta di ripartire le somme complessive sulla base delle quote d'accesso,

che ha spiegato quanto ciascuna Regione ha speso per ogni positivo. La vituperata Lombardia - io non sono lombardo e non sono neanche della Lega Nord, ma di Fratelli d'Italia

Voi togliete il denaro alle Regioni che hanno vissuto l'emergenza e l'aggiungete alle Regioni che l'emergenza non l'hanno neanche vista (quella del *lockdown*; poi forse adesso qualcosa cambierà). cambierà). Francamente tutto ha un limite, tutto può essere opinato rispetto al buon senso. Noi abbiamo preparato due emendamenti, uno sulla scadenza, che abbiamo trasformato in ordine del giorno, e uno sulla famosa tabella. Abbiamo proposto, invece della tabella B,

chi ha riempito le televisioni e i giornali di immagini che tutti noi abbiamo stampate in testa. Questo è un affronto al buon senso. Questo è fare la politica al rovescio e non è possibile che si vada avanti ad oltranza, senza che voi stessi ve ne rendiate conto e senza che facciate appello al vostro buon senso e alla vostra capacità di entrare nel merito dei provvedimenti e di giudicarli.

Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, intervengo molto brevemente proprio per richiamare l'attenzione su un tema che è stato già proposto poco fa dal senatore Floris. Lo faccio con molta amarezza, perché devo constatare che, al di là delle belle parole che sono state dette mille volte in Sardegna, durante le visite di esponenti politici spesso di Governo e di qualunque formazione - anche nel passato, gli impegni che vengono assunti nell'isola regolarmente poi non vengono mantenuti, anzi vengono messi nel dimenticatoio. L'amarezza deriva dal respingimento di un emendamento che avevo presentato, per l'ennesima volta, sulla possibilità di realizzare la rete del metano in Sardegna. Ancora una volta, con motivazioni risibili, che rasentano il ridicolo, e che di fatto celano maldestramente problemi di natura ideologica, quell'emendamento è stato respinto. Cosa deriva da questo fatto? La Sardegna è l'unica Regione nella quale il metano non c'è. non c'è. L'assenza del metano ovviamente porta delle conseguenze gravissime sull'economia della Sardegna, come costi elevatissimi, nettamente superiori a quelli presenti nel resto d'Italia; a questo si assommi la situazione che si vive a causa dell'insularità e del fatto che la continuità territoriale, per incuria, ancora una volta, e per poca attenzione ai problemi dell'isola, non viene applicata. Tutto questo produce produce effetti devastanti sull'economia isolana, soprattutto in questo periodo, che non è soltanto legato all'emergenza Covid-19. Certo, mi disturba leggere su un giornale che, secondo il segretario generale di Hydrogen Europe «l'Italia ha il potenziale per diventare l'*hub* europeo dell'idrogeno nei prossimi decenni perché è dotata della rete di gas più estesa del continente». Ciò significa che ci avviamo ad utilizzare l'energia derivata dall'idrogeno, ma che la Sardegna sarà tagliata fuori anche da questo passaggio perché, in maniera assolutamente incomprensibile, non si consente di realizzare la rete per la distribuzione del metano. È meglio far girare per le strade quelle "bombe" cioè le autobotti contenenti metano che

piuttosto che realizzare una rete che è diventata assolutamente indispensabile. In questo senso mi domando se anche questo Governo si ricordi che la Sardegna fa parte dell'Italia, come tutte le altre Regioni.

Il Governo non ha detto una parola. Io aspetto di vedere delle azioni concrete a tutela della mia isola e che, in qualche maniera, ci si muova perché così non si può andare avanti. Devo dire che in questa circostanza avevo pensato addirittura di non votare la fiducia,

volgere lo sguardo a quest'isola, perché non si può andare avanti in questa maniera. Noi viviamo una condizione di difficoltà estrema: la disoccupazione è alle stelle e non possiamo fare nulla se non cercare di metterci al pari con le altre Regioni, però consentitecelo. Aspetto dei segnali seri nei prossimi provvedimenti, perché è già la terza volta che non si prende in considerazione questo tema che è importantissimo e rilevante per l'economia della Sardegna. Aspetto segnali seri dal Governo e un impegno preciso, perché altrimenti dovrò prendere delle decisioni molto a malincuore. Siccome rappresento il territorio

(e già questo la dice lunga), vorrei parlare, occhi negli occhi, con il vero interlocutore cui ognuno di noi in quest'Assemblea e dai banchi del Governo dovrebbe rivolgersi: i giovani. Il mio intervento oggi è per voi, giovani. Vorrei che foste qui, ora, per sentire la vostra voce e mettendomi nei vostri panni come "diversamente giovane" che non smette di sognare e credere in un mondo migliore che passa, per esempio, da una scuola migliore. A proposito, oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti che, invece di essere al vertice della piramide sociale sono ancora a mendicare concorsi per essere stabilizzati, con dirigenti scolastici ai quali dovremmo fare un monumento per come riescono a supplire

Cari giovani, vi sento e vi ascolto, perché ogni scelta, ogni decisione e ogni linea di indirizzo presa oggi, in questo momento storico così particolare, condizionerà la vostra vita. È arrivato il momento che veniate coinvolti in maniera diretta,

non possono essere solo i pericolosissimi monopattini elettrici senza regole, mentre le bollette aumentano in maniera insostenibile. Non vi è alcun piano concreto e strutturale per combattere il dissesto idrogeologico che distrugge territori e prende vite. Vediamo tutti cosa sta succedendo oggi in Lombardia, Piemonte e Liguria. Cosa vogliamo fare dell'Italia? Un cumulo di macerie? Diamo pure la colpa ai sindaci, non contenti; e per fortuna è passato un nostro emendamento sul reclutamento dei segretari comunali. Giovani, rivendicate il diritto di non dover abbandonare i vostri territori perché magari abitate in montagna o in un piccolo Comune del Salento o della Sicilia; chiedete insieme a noi, a gran voce, le zone a economia speciale per avere sgravi fiscali e semplificazioni per rimanere a casa vostra. Per fortuna, è stata accolta la nostra proposta per promuovere l'imprenditorialità giovanile *under* 30, che consente di guardare al futuro e che deriva da un disegno di legge ancor più composito, a prima firma della senatrice Anna Maria Bernini ma sottoscritto da tutto il Gruppo Forza Italia. non di solo Covid si ammala l'uomo. «Libertà è partecipazione» cantava Gaber, e senza partecipazione saremo costretti a subire le scelte, perché le scelte di oggi determineranno per il nostro Paese, cari giovani, lo stare al di qua o al di là del confine tra essere liberi e protagonisti o essere sudditi. È una linea sottile e il tempo e l'emergenza non giocano a favore. favore. Apriamo una parentesi sull'emergenza. L'emergenza vale quando fa comodo; non vale, per esempio, quando si parla del nemico numero uno in questo momento di crisi economica: le tasse.

con un'Agenzia delle entrate che è forse l'unico ufficio pubblico che funziona e che lavora per l'ordinario. Lo sanno bene i commercialisti e i professionisti che si vedono ridurre o azzerare le poche entrate dalle scadenze fiscali. Questo è un uso politico del Covid. Per fortuna siamo intervenuti a dare una mano a qualche categoria, agli ambulanti, ai termali, mentre altri settori muoiono. Vogliamo parlare della cedolare secca per gli affitti commerciali? Ma dove sta il problema nell'introdurla? Almeno si estenda il credito di imposta. L'ho già detto: questo Governo offre un bicchiere di acqua

Domani non ci saranno medici a sufficienza; domani non ci sarà lavoro per tutti. E invece noi cosa facciamo? Ci rendiamo ridicoli stanziando 50 centesimi a testa per la formazione di casalinghe e «casalinghi» (che oggi è ancora l'accezione di utensile da cucina). Ma allora non si farebbe prima a reintrodurre l'economia domestica a scuola? Cari giovani, rivendicate le pari opportunità contro l'uno vale uno senza senso, valorizzando invece le differenze: il paradigma va invertito. Pari opportunità per tutti non vuol dire livellare tutto verso il basso ma, al contrario, innalzare la possibilità di ognuno dando modo a tutti di accedere ai servizi migliori. Penso alla Regione Lombardia, alla dote scuola, al sistema integrato della sanità; tante state facendo per affossare la Regione marito che... insomma, lo sapete. Senza un progetto, una coppia scoppia; senza progetto, una città diventa un agglomerato di edifici; senza un progetto, una Nazione sopravvive a ruota delle scelte decise per altre ragioni. Cari giovani, fatevi sentire, perché non di solo Covid muore una Nazione.

un debito che vede ben poche riforme strutturali e molte misure temporanee, importanti sì per far fronte all'emergenza, ma poco influenti per dare un vero rilancio al Paese,

Poco di lungimirante e molto «io speriamo che me la cavo». Persino blindarsi dietro le continue richieste di fiducia fa pensare che questo Governo traballi ad ogni occasione di confronto. Una certezza, purtroppo: l'incapacità di dare risposte concrete. Ci sono 420.000 lavoratori che stanno ancora aspettando la cassa integrazione e circa 15.000 le aziende ancora in attesa. Magari il presidente Tridico si occupasse di trovare un sistema di erogazione veloce, com'è stato fatto con l'aumento del suo stipendio. Si vive di incertezza e, purtroppo, il Governo non ascolta le nostre proposte e così non aiuta il Paese. Pensiamo al turismo: sono a rischio 1,3 milioni di lavoratori del settore, che vale il 13 per cento del PIL nazionale e che è stato fra i più colpiti dalla pandemia. Avevamo chiesto contributi a fondo perduto per far fronte alla crisi che è stata subita in maniera massiccia da tutto il comparto e che poche risposte ha avuto. Avevamo chiesto l'ampliamento dell'utilizzo dei *voucher*, sia per il settore turistico che per quello dell'agricoltura: sordi. Pensate a come affronteremo la stagione invernale in montagna: ad ora non conosciamo le intenzioni del Governo sugli impianti di risalita, mentre non sappiamo se ci sarà il flusso di stranieri: ricordo che ci sono località che solitamente lavorano con l'80 per cento di turisti provenienti dall'estero. Senza risposte certe come si possono programmare investimenti e assunzioni? Oltre a mancare la liquidità, mancano pure le risposte in strumenti concreti, ma utili in questo momento per tamponare situazioni di disagio. In una condizione di incertezza i *voucher* non potevano essere considerati uno strumento utile per colmare il *gap* nel momento di necessità? Per generare posti di lavoro non era meglio investire per sostenere le imprese? Siete convinti che il reddito di cittadinanza sia la panacea ai problemi degli italiani? Che sia un *flop* è ormai sotto gli occhi di tutti, se n'è accorto anche il *premier* Conte: il reddito di cittadinanza è una misura assistenzialistica senza progettualità. Non solo i *navigator* non hanno reperito posti di lavoro, ma i Comuni non hanno saputo, soprattutto quelli a guida grillina, avviare progetti utili alla collettività. Ricordiamo il sindaco Appendino, che ha avviato zero progetti su 20.000 percettori di reddito, mentre la Raggi appena 2.500 su 185.000 percettori. Altra grave carenza del Governo: in Commissione bilancio è stato respinto un emendamento per prorogare lo stop delle cartelle esattoriali, così il 16 ottobre 9 milioni di cartelle esattoriali si abbatteranno sui contribuenti con una valanga di pignoramenti. Il ministro Gualtieri rassicura: ci sarà una ripartenza molto graduale; lasciamo perdere. Purtroppo, come già sottolineato da alcuni miei colleghi, in questi giorni stiamo assistendo alla tragedia del maltempo ed esprimo cordoglio per le vittime e vicinanza ai territori. Avevamo presentato un emendamento per istituire un fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020. È stato considerato troppo oneroso; lo abbiamo trasformato in ordine del giorno e speriamo che non finisca nel dimenticatoio. Ad oggi, mentre la nostra Italia è nuovamente ferita, il ministro Costa scarica la responsabilità sui Comuni per la difficoltà di individuare le zone a rischio e progettare la carenza di risorse, come se le risorse e la burocrazia non dipendessero anche dal Governo centrale. Pensate che, secondo gli ultimi dati del rapporto nazionale sulla situazione del dissesto idrogeologico nel nostro Paese, è a rischio il 91 per cento dei Comuni italiani, con 7 milioni di residenti in zone vulnerabili e non si è stanziato nemmeno un centesimo. Manca una politica chiara, che metta al centro dell'agenda politica interventi per arginare il dissesto idrogeologico e risolvere i problemi legati al nostro fragile territorio. È ora di finirla di scaricare la propria incompetenza su Regioni, Province e Comuni. Questa è un'abitudine di matrice grillina. Prima c'è stata l'Azzolina, che ha riversato sui dirigenti scolastici e sui Comuni l'incapacità di far ripartire le scuole e ora anche il ministro Costa segue questa scia. Meno teorie e più fatti, meno monopattini e più soldi per controllare ponti e ripulire fiumi; meno vincoli e più fondi ai Comuni, subito. A questa maggioranza, sorda alle esigenze di imprese e privati cittadini, diciamo che non si risolvono i problemi facendosi belli e scaricando le responsabilità sugli altri.

alla domanda se questo decreto-legge potesse essere ancora migliorato, la risposta non può che essere ovviamente «sì, certo», e diciamo che in parte è stato migliorato grazie all'azione emendativa delle forze di opposizione e di maggioranza e qualche ritocco è stato fatto anche dal Governo. Governo. Certo che poteva essere migliorato, ma questo Parlamento - quindi noi, ogni singolo senatore - ha la responsabilità

che ha scosso gli equilibri e le economie mondiali, ha turbato e perturbato gli ordinari equilibri familiari, la vita delle persone, delle bambine, dei bambini, degli adolescenti, di donne, uomini, nonne e nonni. Questi comportamenti hanno influito sulla parte sociale del Paese e del mondo e hanno influito notevolmente sulla capacità di reazione che ogni singola economia nazionale poteva e può attivare. Ma questa maggioranza una visione ce l'ha? Qualcuno o qualcuna - penso al Presidente del Senato ha ricordato al Paese che questa maggioranza non ha una visione. Ebbene, io le voglio ricordare che, grazie a questa maggioranza, una visione fortunatamente c'è nel Paese. Abbiamo visto lungo quando abbiamo capito che il Governo giallo-verde aveva collocato il nostro Paese in un angolo del respiro internazionale internazionale e della collocazione europea. Questo significa che oggi abbiamo la possibilità - altro che il gioco dell'oca - di capire quali sono le risorse che possono essere utilizzate nel nostro Paese; se non avessimo avuto la visione non ci sarebbe stato nemmeno questo sogno. Tradotto in parole semplici: senza le risorse europee non avremmo avuto nemmeno la speranza di ritornare

Che cosa abbiamo fatto con questi 100 miliardi? Che cosa hanno voluto fare la maggioranza e il Governo con questi 100 miliardi? Come dicevo prima, non hanno voluto trascurare la coesione sociale la coesione territoriale, nel cuore della pandemia, per difendere la capacità produttiva del nostro Paese dalle conseguenze economiche dell'emergenza, guardando al futuro della nostra economia nello scenario globale. globale. Sulla direttrice di questi decreti che abbiamo inanellato (altro che vivere alla giornata) è stato dato un sostegno al nostro Sistema sanitario nazionale,

prorogate le misure a sostegno dei lavoratori, prolungando ancora per diciotto settimane la cassa integrazione nelle diverse tipologie. E ancora: sgravi contributivi per le aree svantaggiate, oltre a specifiche indennità sui settori ormai in ginocchio e incentivi per assunzioni a tempo indeterminato; rifinanziamento con 7,8 miliardi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; prorogata la moratoria sui prestiti e mutui; 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato; Fondo emergenza cinema, spettacolo e audiovisivo; 200 milioni per potenziare l'attività di trasporto, tra cui taxi, NCC, autotrasporto, autobus turistici e servizio viaggiatori e crociere. Tante le misure in campo fiscale: risorse ingenti destinate a Comuni, Città metropolitane e Regioni per fronteggiare le minori entrate. Potrei continuare nell'inanellare le misure e gli interventi previsti da questo decreto-legge. passerà dalla capacità che avremo nella realizzazione di progetti di rilancio del Paese, utilizzando tutte le risorse che l'Europa ci mette a disposizione, a partire dalle risorse del MES, perché se è vero che il nostro Paese era già in difficoltà nel comparto sanitario e abbiamo la necessità di intervenire, servono delle risorse. E se non dovessimo reperire le risorse dalla voce europea, dobbiamo liberare quelle risorse da altre voci e da altri comparti oggi già in difficoltà. Sono sicuro che su questo, anche su questo, la maggioranza saprà trovare una sintesi per rilanciare al meglio il nostro Paese e la nostra economia. Riprendo un concetto che ho voluto condividere in Commissione lavoro, che è stato ripreso brillantemente dalla collega Fedeli, sul rapporto tra sicurezza del lavoro, sicurezza sociale, investimento sul capitale umano e crescita: vanno di pari passo. Oggi con il Covid è cambiato completamente il mondo: *ante* parlavamo di salario minimo; oggi dobbiamo spiegare che un conto è la giusta retribuzione (e su questo ci affidiamo alla contrattazione collettiva

la violazione del diritto umano. Quindi dobbiamo trovare due livelli: uno è la giusta retribuzione e l'altro è un livello al di sotto del quale nessuno può portarsi.

all'articolo 27 sulla coesione territoriale, recante agevolazioni contributive per l'occupazione in aree svantaggiate e decontribuzione al Sud. Su questo tema purtroppo esprimo una nota di amarezza, perché anch'io ho presentato un emendamento e la pongo come questione politica importante. Infatti, lo stesso approccio che ha visto correttamente l'investimento e l'attenzione per una coesione territoriale per le aree del Sud deve essere attivato per le aree metropolitane e per le zone in difficoltà, perché non sono sufficienti le lucine di Natale per attivare le aree di crisi Noi abbiamo la necessità - il mio emendamento lo prevedeva - di intervenire favorendo micro e piccole imprese, attivando delle zone franche. Zone franche significa burocrazia zero e e fisco zero e questo lo si può fare con ragionevolezza. Solo ed esclusivamente con questa tipologia di intervento e con questo approccio possiamo risollevare le sorti delle aree metropolitane depresse che vanno dal Nord al profondo Sud. Pongo questa come una questione politica.

del Consiglio su quelle che potrebbero essere le eventuali ulteriori restrizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica. Quindi siamo in un momento critico

In molti casi, quindi, i provvedimenti deliberati, votati in quest'Aula, votati dal Parlamento, sono rimasti assolutamente lettera morta. Questo è un problema gravissimo

comunicazione che fa il Governo e il Paese reale. Il Governo comunica provvedimenti roboanti, provvedimenti bazooka e invece il Paese reale è un altro. Ancora una volta ci ritroviamo a parlare della distanza che c'è tra la comunicazione del Governo e la realtà.

solo provvedimento che prevedesse norme chiare da scrivere tutti quanti insieme. Invece, molti colleghi della maggioranza ci hanno persino deriso su questi 100 miliardi. Oggi siamo arrivati a 100 miliardi, ma con tanti piccoli provvedimenti spezzatino che non stanno portando e producendo effetti positivi per

dopo vorrei ricordare alcune cose. Non si genera oggi consumo parcellizzando in questo modo la spesa o mettendo a disposizione questi *bonus*. Anzi, gli effetti sono doppi e negativi perché i *bonus* hanno una quantità

che abbiamo definito assistenzialistiche e che non servono assolutamente in questo momento al rilancio del nostro Paese per sostenere gli investimenti.

che ci aspettano saranno importanti e decisive. Il Governo sarà chiamato alla sfida più importante degli ultimi anni, la seconda sfida storica più importante dopo quella del dopoguerra. Il Governo sarà chiamato all'impegno europeo importante di elaborare proposte, progetti e riforme. Del cosiddetto *recovery fund* ne abbiamo parlato in tanti e lo stiamo studiando tutti, però, come dicevo, è il Governo che deve dare

politici e tecnici, perché se non ha funzionato su questi provvedimenti, ahimé sarà difficile che possa funzionare su un provvedimento e su una sfida importante

di riuscire a trovare delle soluzioni, di essere snelli e soprattutto di guardare al futuro. Per questo vorrei concludere, signor Presidente, parafrasando Seneca che diceva che nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

decreto agosto si inserisce in perfetta linea di continuità con il decreto cura Italia e con il decreto rilancio. Il sostegno all'economia e gli incentivi per la ripresa piena dei consumi sono obiettivi di lunga prospettiva e richiedono interventi costanti e coerenti. In tale ottica va osservato il pacchetto di norme che il Governo ha presentato alle Camere. Se è vero che le difficoltà che stiamo affrontando nel 2020 sono straordinarie, è altrettanto vero che straordinarie sono le risposte del nostro Governo. Il supporto alla crescita, ai lavoratori, agli imprenditori e alle famiglie è quantificabile economicamente ed è sotto gli occhi di tutti. Ammontano infatti a 100 miliardi di euro le risorse totali che lo Stato ha messo in campo con i provvedimenti adottati fino a questo momento, grazie anche all'ulteriore scostamento di bilancio approvato dal Parlamento. Di questi, ben 25 miliardi rappresentano le ulteriori somme che con il decreto agosto andranno a produrre effetti positivi su tutto il Paese; un'occasione storica, anche grazie al successo del Presidente del Consiglio nella negoziazione europea, che ha permesso l'utilizzo molto più espansivo della politica fiscale. Per questo si può affermare che che siamo davanti ad un *new deal* italiano ed europeo che permetterà al Paese di avere la ripresa che merita. Il percorso iniziato e perseguito dal Governo con il decreto agosto reca misure innovative e di sviluppo, mettendo in campo proposte di fiscalità agevolata, incentivi a fondo perduto, di finanziamento di strumenti a supporto delle imprese, nonché nuove indennità per i lavoratori che più hanno subito gli effetti del Covid-19. altro, però, porta con sé un nuovo approccio sistemico alla questione meridionale, che da troppo tempo affatica l'economia italiana, non permettendone il pieno sviluppo. Per la prima volta, infatti, il Governo approva uno strumento pensato per colmare il divario tra le Regioni del Sud e quelle del Nord; divario che inevitabilmente si ripercuote sui cittadini, sulle loro possibilità e ambizioni e sulle infrastrutture di cui potrebbero usufruire. L'argomento mi è molto caro, non solo per la mia provenienza, ma anche e soprattutto perché credo convintamente che annullare le differenze territoriali sia l'unica via per poter superare la crisi economica. Riprendendo le parole del presidente Conte, sono certa che il decreto agosto ponga le basi per un processo di reindustrializzazione del Sud, possa essere cioè un volano per l'economia e un'attrattiva per le aziende che vogliono investire nel Meridione. In concreto, le misure previste permettono di incidere in modo non non trascurabile su circa 500.000 imprese, delle quali oltre il 90 per cento ha meno di dieci dipendenti. Si tratta, dunque, di piccole e medie realtà imprenditoriali che costituiscono lo zoccolo duro dell'economia italiana. Nello specifico, quello che stiamo realizzando è un abbattimento del costo del lavoro per tutti i lavoratori dipendenti, con una fiscalità di vantaggio che prevede una decontribuzione per l'impresa pari al 30 per cento delle imposte sul lavoro dipendente, a partire dagli inizi di ottobre fino a dicembre 2020 e che mi auguro verrà riconfermata con la prossima legge di bilancio. A questo si aggiunge un'attenzione generale per il settore del lavoro, sul quale ricadono le misure a mio parere più incisive del decreto-legge. Ricordo, a titolo esemplificativo, il rifinanziamento della cassa integrazione per ulteriori diciotto settimane, al quale si affianca la possibilità per gli imprenditori di far rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione e giovare, in alternativa, di uno sgravio contributivo del 100 per cento per In tal modo siamo sicuri di garantire sostegno all'occupazione e alle imprese che si trovano maggiormente in difficoltà. Inoltre, nel campo delle politiche attive del lavoro e della formazione, il decreto-legge prevede il finanziamento di 500 milioni - per il biennio 2020-2021

sia per le imprese che godranno di dipendenti più specializzati sia per gli stessi lavoratori che godranno di una maggiore preparazione, che permetterà loro - ove necessario - di transitare verso altri impieghi aumentandone la possibilità di occupazione. Siamo inoltre davanti a un provvedimento che garantisce una spinta all'occupazione, prevedendo una decontribuzione del 100 per cento per sei mesi per le assunzioni di nuovi dipendenti a tempo indeterminato, nonché una decontribuzione del 100 per cento per tre mesi del lavoro stagionale Questo settore è tra i più martoriati dall'epidemia Covid-19 e anche tra i più interessati dalle risorse del decreto-legge agosto. Con tale provvedimento abbiamo infatti confermato l'indennità ai lavoratori del settore del turismo e delle terme. Vorrei ricordare che per garantire liquidità alle imprese sono stati contestualmente rifinanziati alcuni strumenti di supporto. Tra questi, ricordo i 64 milioni per la nuova Sabatini, i 500 milioni per i contratti di sviluppo e i 950 milioni per il fondo per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo. Ancora, abbiamo rifinanziato per 7,8 miliardi di euro, per per il triennio 2023-2025, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese allo scopo di favorirne l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. In tema di piccole e medie imprese ricordo anche la moratoria sui prestiti e sui mutui fino al 31 gennaio 2021 nonché gli incrementi previsti per i fondi legati al mondo della cultura e dello spettacolo, che hanno gravemente subito gli effetti della pandemia. Queste sono solo alcune delle misure pensate e attuate per fronteggiare la crisi e riorganizzare la ripartenza, alle quali si aggiungono incrementi di notevoli fondi istituiti dal decreto-legge dal decreto-legge rilancio, come, ad esempio, il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, nella consapevolezza che per poter attuare appieno il principio di sussidiarietà nel superamento delle enormi difficoltà che la pandemia ci ha messo davanti è necessario garantire agli enti locali e alle Regioni le risorse sufficienti. Tutto questo e molto altro è contenuto nel decreto-legge agosto, che è un pacchetto vasto e con amplissimo respiro, il quale, coinvolgendo molti settori diversi, cerca di non dimenticare nessuno. Per queste ragioni, a chi dai banchi dell'opposizione continua a ripetere stancamente e strumentalmente che troppo poco è stato fatto, mi permetto di ribattere prendendo in prestito le parole del poeta greco Esiodo: «Se aggiungi poco al poco,

esame introduce ulteriori misure, volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia le risorse impiegate a tal fine sono in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento, autorizzato con ben due risoluzioni,

non sia corretto avere questo tipo di atteggiamento. Certo, si fa il gioco delle parti, per carità di Dio, ma non è corretto nei confronti dei relatori, che davvero hanno accolto tutte le istanze e hanno ascoltato tutte le esigenze, che venivano anche dalla minoranza.

questa Agenzia, punto di raccolta di dati fra l'Agenzia e lo Stato (il Ministero della salute) e le Regioni. Sono dati importanti, che non risolveranno il problema - certo che no: avremo ancora le liste d'attesa

riconosciuto che il nostro Paese sta andando meglio rispetto agli altri, perché questi provvedimenti - che tutti stanno criticando - hanno comunque portato a un miglioramento e a una positività: abbiamo un modello che possiamo perseguire e, anzi, facciamo scuola anche agli altri Paesi. *(Applausi)*.

Mi sembra che lo stiamo riducendo a qualcosa di diverso da quanto delineato dalla Costituzione. La nostra Costituzione mette al centro di tutta l'azione politica e dello Stato il Parlamento. Ma come è possibile che non ci sia stata più nessuna valutazione? Ora la collega Boldrini si chiedeva perché ci sia stata una lunga discussione in Commissione, ma non si chiede

di partito, ma di studio del diritto e della Costituzione. La stessa origine ci ha portato a fare forse la stessa riflessione.

quattro giorni fa - che vi è un pericolo per la democrazia parlamentare nel momento in cui si susseguono decreti-legge convertiti tutti con la fiducia. Questa è una questione

Badate, non è che lo diciamo oggi. Senatore Mirabelli, quando ero Sottosegretario mi sono sempre opposto a riunioni di maggioranza, perché ho sempre ritenuto necessario coinvolgere l'opposizione. Perché va coinvolta l'opposizione? Forse per garantire all'opposizione una partecipazione alle decisioni? No,

di credito e di avere dei finanziamenti. Questa è la vostra capacità di crescita. Nello stesso tempo, dal 15 ottobre era prevista la proroga della riscossione coattiva delle imposte e da quella data scatterà la nuova riscossione coattiva. Signor Presidente, se fossi un po' populista, come alcuni presenti in questo Parlamento, dovrei dire che forse non è più il caso di fare stampe di questo tipo per ogni decreto-legge convertito con la fiducia, perché nessuno di noi riesce a leggerle.

si avesse cognizione, non ci troveremmo nella situazione che ho appena denunciato, quantomeno per le aziende. Noi avremmo avuto necessità di uno sviluppo complessivo del sistema produttivo del nostro Paese, perché questo serviva per garantire

secondo questo sistema, ossia con un decreto-legge convertito con la fiducia, ma con una concertazione precedente all'ingresso in Parlamento, perché il Parlamento servirà soltanto ad approfondire le questioni che eventualmente il Governo, sentendo l'opposizione...

chi mi ha preceduto ha già parlato ampiamente del contenuto del provvedimento in esame, toccando articoli e facendo riferimento per l'ennesima volta

in tutti i suoi segmenti e ha praticamente inciso molto su ogni parte sociale. Il senatore Laus ha anche aggiunto che c'è comunque una visione di questa maggioranza. A me spiace doverlo ripetere,

dei colleghi senatori di minoranza, che rappresentano pur sempre una fetta abbastanza copiosa degli italiani:

vi hanno fatto presente quali articoli sono solo "spizzichi e mozzichi" rispetto alle reali esigenze. Invece

Il ministro Costa, visto che è su tutti i giornali il disastro idrogeologico che sta avvenendo in più Regioni, fa riferimento al fatto che è molto ottimista perché i fondi ci sono: ci sono: 7 miliardi sono in cassa. Ma c'è un problema piccolo, una cosa da niente: mi riferisco al decreto semplificazioni che sicuramente romperà tutti i lacci e lacciuoli di natura amministrativa e burocratica.

la vergogna, perché un conto è andare di fretta, spicciarsi, muovere, semplificare e sburocratizzare; un conto invece è arrivare di corsa e dover ricorrere alla fiducia con un provvedimento che, analizzato bene,

Le riforme hanno bisogno di contenuti e i contenuti devono avere un valore talmente pesante da giustificare l'uscita di oltre 100 miliardi, che si aggiungono

qua dentro, in una procedura semplificata, veloce, senza lacci e lacciuoli, si siano affidati a una ditta di Cerignola, la Cerichem Biopharm,

per 12.000 euro, per 25.000 litri di gel disinfettante; un terzo accordo per 21.000 euro, per 5.000 confezioni di salviettine, 50 *spray* disinfettanti, 170 visiere

all'interno, direttamente con l'Esecutivo, e poi, quando è ora di semplificare una norma che dà la possibilità a quelli che fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, ci si rifà alla paura che i cittadini possano delinquere.

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il decreto agosto si inserisce in perfetta continuità con il decreto cura Italia e con il decreto rilancio e - non a caso - il provvedimento che stiamo trattando oggi è anche chiamato il decreto rilancio 2, sebbene introduca numerosi elementi di novità. Lo spirito del provvedimento, come i due precedenti citati, è continuare a estendere e rafforzare la rete di protezione attorno ai nostri imprenditori, al nostro tessuto economico-produttivo, messo a dura prova dalla pandemia da Covid-19, e a porre le condizioni per rilanciare la nostra economia combinando misure di aiuto temporaneo e misure di prospettiva, che guardano al futuro e allo sviluppo economico.

e i 55 del decreto rilancio, il decreto agosto fa arrivare a 100 miliardi di euro la mole di risorse messe in campo per far fronte alla emergenza Covid. Tante sono le misure di aiuto a sostegno confermate e prorogate: su tutte cito la proroga della cassa integrazione in deroga e il rifinanziamento per gli anni a venire del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese con più di 7 miliardi di euro. Numerose sono le nuove misure di sostegno ai lavoratori e operatori economici, come - ad esempio - l'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi, l'indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo; il sussidio di 600 euro per i lavoratori del settore dello sport; l'introduzione di un fondo per la filiera della ristorazione, con 600 milioni di euro per il 2020, per garantire contributi a fondo perduto per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, con l'obiettivo di valorizzare le produzioni locali. cito l'introduzione di contributi a fondo perduto per i negozi dei centri storici, che sono stati penalizzati dal calo dei flussi turistici sempre in conseguenza della pandemia; contributi che non saranno inferiori ai 1.000 euro per le persone fisiche fisiche e ai 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e fino a un massimo di ben 150.000 euro. Numerose e corpose sono le misure che guardano al futuro e allo sviluppo sostenibile e tecnologico: abbiamo infatti stanziato 500 milioni aggiuntivi per il fondo nuove competenze per la formazione dei lavoratori; abbiamo incrementato di 500 milioni di euro per il 2021 le risorse assegnate ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Abbiamo incrementato di 500 milioni per il 2020 le risorse per i contratti di sviluppo; abbiamo potenziato di 950 milioni per il 2021 la dotazione finanziaria del fondo IPCEI per l'attuazione dei progetti di comune interesse europeo nel campo della ricerca, sono anche le proroghe fiscali per dare ossigeno al nostro tessuto economico e produttivo: abbiamo introdotto la possibilità di rateizzare ulteriormente almeno il 50 per cento del valore dei versamenti fiscali precedentemente sospesi e questa rateizzazione si estenderà estenderà per buona parte del 2021; abbiamo prorogato al 20 aprile 2021 il termine di pagamento del secondo acconto dell'imposta sui redditi o dell'IRAP per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, il cosiddetto ISA. Abbiamo prorogato dal 31 agosto al 15 ottobre il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento o avvisi esecutivi. Durante l'*iter* parlamentare di questo decreto-legge sono stati introdotti diversi miglioramenti: per esempio è stato prorogato al 30 ottobre il termine dei versamenti d'imposta per i contribuenti per i contribuenti sottoposti agli ISA. È stato prorogato al 15 ottobre l'esonero dal pagamento della TOSAP per gli ambulanti, che è una misura aggiuntiva rispetto a quella che prevedeva l'esonero fino al 31 dicembre per bar e ristoranti. Per ciò che riguarda poi il superbonus del 110 per cento, è stato reso più chiaro il percorso di asseverazione che dovranno fare i tecnici e i progettisti e sono state abbassate le soglie di deliberazione dei condomini per accedere al finanziamento bancario o allo sconto in fattura o per cedere il credito d'imposta agli organismi finanziari. È stato reso più chiaro il concetto di accesso autonomo all'edificio: tutte misure che tendono a facilitare e ampliare la platea dei beneficiari. Sono state poi potenziate le tutele nei confronti dei lavoratori fragili, prevedendo che fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati tali - a solo titolo di esempio: i malati oncologici, gli immunodepressi, i disabili di cui alla legge n. 104, eccetera eccetera - il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e dopo questa data potranno utilizzare lo *smart working* fino a fine anno. E questi sono appunto solo alcuni esempi. Presidente, al di là delle polemiche e polemichette strumentali e propagandistiche, è impossibile non vedere la quantità e la qualità dello sforzo profuso per combinare protezione dei cittadini e delle imprese e rilancio del Paese. Fa specie che le critiche provengano proprio da coloro - e mi riferisco alle forze politiche che sostenevano il Governo del centrodestra - che, durante la crisi originata nel 2008 e che è andata avanti poi per molti anni, non hanno mosso un solo dito, nemmeno un dito, assistito inermi alla sparizione di quasi 500.000 imprese e di centinaia di migliaia di posti di lavoro. E ora ci vengono a fare la morale e la lezioncina! Non va dimenticato, Presidente, che si avvicinano la stesura e l'esame della legge di bilancio, che metterà a disposizione risorse aggiuntive, tra i 30 e i 40 miliardi di euro, e che negli auspici dovrà essere concepita in combinato disposto con il *recovery fund*. con il *recovery fund*. Alcune importanti misure per il nostro sviluppo futuro potranno poggiare su impegni di spesa finanziati nel corso del 2021 dai fondi *recovery*. Tutto questo ci consentirà di concentrare gli sforzi su altri obiettivi importanti per il Paese, sui quali il MoVimento 5 Stelle ha lavorato incessantemente e lavorerà ancora. Mi riferisco alla stabilizzazione del superbonus del 110 per cento, quindi oltre il 2021; alla stabilizzazione dei consistenti incentivi per le imprese del piano transizione 4.0, che - lo ricordo - già oggi valgono sette miliardi di euro l'anno; alla proroga della decontribuzione decontribuzione al 30 per cento per le imprese del Sud, che è una misura importantissima introdotta dal decreto agosto, e quindi da questa maggioranza e da questo Governo, che sarà vitale prorogare vista l'importanza per il Paese che rivestono il rilancio e la ripresa del Sud. Nella stessa legge di bilancio si porranno le basi per una organica riforma dell'Irpef, che non potrà prescindere da un drastico alleggerimento della pressione fiscale e delle spese sul ceto medio, preceduta però da due misure immediate, e cioè la conferma del taglio del cuneo fiscale per 16 milioni di contribuenti, già approvata da questo Governo per il secondo semestre del 2020, e il debutto dell'assegno unico per i figli, che agevolerà la vita delle famiglie razionalizzando la giungla dei *bonus* oggi esistenti. In conclusione, il MoVimento 5 Stelle continuerà a lavorare senza sosta per dare ogni possibile sollievo ai cittadini e per mettere l'Italia sul percorso del rilancio che merita. Per questo sarà decisiva la spesa degli ingenti fondi *recovery* ed è un risultato storico, questo, che è stato conseguito in Europa ed è dovuto anche al nostro costante stimolo. Su questo non ci siamo mai fermati. *(Applausi)*.

evidente a tutti come questa maggioranza e il suo Governo abbiano finito anche la fantasia. Fino ad oggi almeno quella non vi mancava: il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, il decreto cura, il decreto liquidità, il decreto rilancio. Ad un certo punto vi siete accorti anche voi che avevate esaurito persino la fantasia delle denominazioni

la mancanza di una politica per affrontare la grave crisi e dare un senso all'indebitamento dello Stato che avete realizzato; un indebitamento, questo sì, senza precedenti. Le decine di miliardi che snocciolate ad ogni passo, elencando un miliardo per questo, cento milioni per questo, cinque milioni per quest'altro, partono da un presupposto che non ammettete mai: non si tratta di un tesoro che avete trovato sotto l'albero; non sono risorse che avete creato grazie a una politica fiscale o a una politica produttiva che abbia portato a nuove entrate. I 100 miliardi di cui parliamo sono 100 miliardi di nuovo indebitamento dello Stato con tre scostamenti di bilancio; 100 miliardi che nessuno ha mai avuto per realizzare una manovra in questo Paese, 100 miliardi che

100 miliardi in più e di quelli che vi apprestate a elencare con il *recovery fund* o con altre misure europee. È come se aveste trovato un tesoretto a Roma e poi, improvvisamente, un altro più importante tesoro a Bruxelles. Non è così

ancora deciso come realizzare. Ove non fosse realizzata la tassazione sul digitale o sulla transazione finanziaria, sarebbe sempre parte del nostro bilancio per la parte che ci compete. E se ciò dovesse avvenire, sventuratamente, alla fine, dei 209 miliardi il guadagno italiano a fondo perduto sarebbe di 25 miliardi. Il resto - parliamo di centinaia di miliardi:

Chi ha visto qualche risultato di questi 100 miliardi? La vostra manovra è tutta fatta di mance e di micro provvedimenti.

intervengono ben dodici Ministri, ciascuno con le sue piccole cose, ma non emergono una strategia

Abbiamo suggerito negli emendamenti presentati di creare una sorta di compensazione fiscale con quanto le imprese hanno già versato come anticipo fiscale nel novembre dello scorso anno per IRAP e Irpef. Almeno diamo direttamente alle imprese che ne hanno bisogno bisogno e hanno già pagato il fisco; alle imprese attive che, comunque, contribuiscono al benessere del nostro Paese e alle entrate fiscali. Attraverso compensazioni fiscali evitiamo di lasciarle nelle mani di nessuno e di disperdere i *bonus* a pioggia che nessuno realizza. Tutti i nodi industriali del Paese sono ancora lì a dover essere risolti, e ne elenco alcuni che costituiscono anche le vostre battaglie: non sappiamo e e non sapete nulla - questo è ancora più grave - di come finirà la vertenza su Atlantia, con il titolo che fa balzi in borsa a ogni dichiarazione. Chissà quando indagheranno su quelle dichiarazioni e sulle conseguenze della borsa e sui titoli azionari di Atlantia. Lo dico al movimento della trasparenza. della trasparenza. Non sappiamo e non sapete nulla del destino dell'Ilva e del settore siderurgico. Non sapete cosa accadrà perché non lo avete ancora stabilito, ove si ritirasse il colosso indiano. sapete che la bandiera di Whirlpool chiuderà e con essa chiuderanno molte delle centinaia di imprese ai tavoli di crisi del Ministero.

conosciamo tutti quanto accadrà se entreranno in vigore - ed entreranno in vigore - le nuove regole sulla collocazione del debito delle imprese e dei cittadini, la gran parte dei quali finiranno tra gli insolventi. Questa montagna, questo macigno, questa bomba atomica rischia di destrutturare il sistema produttivo e sociale italiano. Di questo vorremmo che voi parlaste. E, soprattutto, vorremmo che un Governo serio, dotato di una strategia e di una visione, intervenisse prima che - da una parte - l'enormità del debito pubblico che si sta accumulando parte - la bomba atomica dei crediti deteriorati, che dovrebbe disossare il tessuto sociale e produttivo del Paese, possano piegare davvero la Nazione italiana. Non lo permetteremo.

contiene importantissime e ingenti risorse che vanno a contribuire, dopo altri provvedimenti, a dare sostegno al nostro Paese. Mi riferisco ai 25 miliardi che fanno seguito agli importanti stanziamenti del precedente decreto-legge cura Italia, del decreto rilancio, oltre alle misure del decreto semplificazioni. Sono state importanti, anche in questa occasione, le misure messe in piazza dal Governo sui temi del lavoro, su questioni fiscali,

con specifici emendamenti ha apportato numerosi miglioramenti in diversi ambiti e settori. Brevemente vorrei ripercorrere alcuni passaggi che sono frutto del lavoro del Gruppo Italia Viva-P.S.I., che spesso hanno trovato

alla proroga di una serie di versamenti per quei professionisti, per quelle realtà che applicano gli indici sintetici di affidabilità;

sulle donne; agli emendamenti legati al mondo della disabilità, con la continuità didattica per il sostegno scolastico ai ragazzi necessitanti di questo tipo di supporto e sostegno; allo *smart working* per i genitori di persone con disabilità grave riconosciuta; al *bonus* ristoratori, esteso ad agriturismi con ristorazione, catering per eventi e ristoranti degli alberghi. Allo stesso modo, le misure del terremoto hanno messo insieme proposte e suggerimenti provenienti da diversi colleghi. l'aiuto ai lavoratori fragili: un'importantissima misura per le ingenti risorse che il Senato ha utilizzato tra quelle a disposizione, integrandole al contempo grazie a uno sforzo straordinario da parte del Governo, che va incontro ai bisogni di chi, per ragioni di salute, si trova in condizioni di grave difficoltà nel riprendere il proprio lavoro e la propria attività. Ancora, vi sono: il fondo prima casa; la proroga all'avvio dei lavori di efficientamento energetico per i Comuni, spostando in là le scadenze che la legge di bilancio aveva previsto; la misura che finalmente toglie - anche nel nostro Paese - l'obbligo di utilizzare solo fino a un massimo del 50 per cento plastica riciclata

fino ad un massimo del 100 per cento di platica riciclata utilizzabile - il *tax credit* per gli spettacoli dal vivo; la rivalutazione dei beni anche per quei soggetti che hanno un bilancio d'esercizio che non coincide con l'anno solare. Insomma, abbiamo dato un contributo importante, come tanti colleghi di altri Gruppi, al miglioramento del decreto-legge Ora, però, abbiamo lo sguardo che già volge - da un lato - verso la legge di bilancio e - dall'altro - verso gli importanti provvedimenti che dovranno essere presi grazie all'utilizzo delle risorse del *recovery fund*. il Governo anzitutto - con le proposte che elaborerà - ma anche il Parlamento, il Senato in modo specifico, con il proprio potere di indirizzo nei confronti dell'Esecutivo, dovranno dare all'utilizzo di queste risorse ingenti una finalizzazione strategica. Non dobbiamo correre il rischio di usare le risorse a pioggia, cercando di coprire tante richieste ed esigenze che arrivano da ogni parte, non solo da settori produttivi, da filiere, ma anche da altre istituzioni, dalle Regioni, dagli stessi Credo che ogni realtà locale ambisca a poter utilizzare parte di queste risorse per qualcosa di specifico, magari di mai risolto nel passato, ma, badate, cari colleghi: non dobbiamo cadere proprio nella tentazione di di distribuire a pioggia le risorse laddove magari non si è riusciti nel tempo e negli anni ad arrivare con le misure delle leggi di bilancio o magari anche con quelle previste nei decreti-legge che abbiamo approvato approvato in questo anno. Abbiamo il dovere di concentrare le risorse ove servono per cambiare passo al nostro Paese, per cambiare l'Italia ove è necessario farlo; per raggiungere quelle zone del Paese che non sono ancora servite da infrastrutture importanti, dall'alta velocità. Il collega Cucca prima ricordava la metanizzazione della Sardegna: uno scandalo che ancora un'intera Regione non abbia un servizio come questo, quando il Paese intero è annoverato in Europa tra quelli con una maggiore rete di metanizzazione. Serve arrivare non alle piccole cose, ma alle operazioni che possono cambiare il volto del Paese. Il tema della cultura, che è identità, che è alla base della stessa conoscenza del nostro Paese nel mondo, credo dovrà essere uno degli ambiti sui quali si dovrà investire maggiormente per fare ancora di più attrazione di tipo turistico per il nostro territorio, consentendo in tal modo di sviluppare

L'Italia riesce a sviluppare progetti significativi importanti, ma non così tanti quanto il genio italiano consentirebbe di fare, se si investisse di più. le prossime risorse che dobbiamo ripartire, anche con gli indirizzi specifici che il Parlamento vorrà dare al Governo, dovranno essere indirizzate proprio in questa

sulle modalità e sull'operatività che il Parlamento ha avuto anche in questa occasione, con un ritmo di lavoro che non permetterà alla Camera dei deputati di vagliare pienamente il

per decidere come procedere. Se c'è la necessità di fare modifiche alla Costituzione, perché si arrivi a una diversa modalità di gestione del processo legislativo, credo che sia questo il momento di farlo. Dopo l'esito del *referendum*, le forze politiche che siedono in Parlamento devono interrogarsi - maggioranza e opposizione insieme, possibilmente - su quali misure di cambiamento della nostra Costituzione è necessario approvare, perché lo stile, l'*iter* e la prassi che ormai da diverso tempo prevalgono non sono accettabili. Credo che anche da parte del Presidente della Repubblica ci sia da attendersi un appello, perché con responsabilità si arrivi alle modifiche necessarie per far sì che la nostra Costituzione sia pienamente attuata.

quando nel nostro Paese c'erano temperature con picchi di 30 gradi e il Parlamento si trova a convertirlo oggi, quando sulla nostra penisola inizia ad arrivare l'autunno e alcuni fenomeni di maltempo eccezionale hanno iniziato a colpire i territori, con violenza inaudita. È il caso del Piemonte: citando la mia Regione, mi sia concesso di esprimere in questa sede la massima vicinanza alle famiglie delle vittime del maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Nord Ovest del Paese. Su questo tema sarà necessario intervenire in modo strutturale, partendo dalle infrastrutture e da tutte quelle opere di manutenzione del territorio che non possono più aspettare. È necessario intervenire e farlo presto, a partire dalle risorse del *recovery fund* e senza muovere accuse ai livelli di governo più bassi, come fa oggi sui giornali il ministro Costa, in modo scomposto e poco appropriato. Un Governo che riscontri carenze di competenze nei Comuni più piccoli e in quelli delle aree interne, che sono la spina dorsale del Paese, non può limitarsi ad accusarli, ma deve creare le condizioni, anche in un'ottica sussidiaria,

lo è stata ancora di più durante questa lunga emergenza epidemiologica. Dobbiamo però tornare a dare centralità al Parlamento. Oggi prendiamo atto del fatto che anche questa volta si sia scelto di porre la fiducia. Prendiamo atto del ruolo sempre più marginale che viene lasciato al lavoro delle Camere. Quello che però dobbiamo ancora una volta evidenziare è che in questo provvedimento il Governo prova a mettere toppe su tutto. Lo stesso viene peraltro fatto con le linee guida del piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo dunque di fronte a un *modus operandi* di questo Esecutivo: si prova intervenire su tutto, senza un piano strategico, e questo modo di non guidare il Paese è molto preoccupante. La parte migliore del Paese, però, non chiede non chiede assistenzialismo, ma interventi e opportunità da declinare in modo strutturale nel lungo periodo e risposte concrete alle necessità stringenti. Su questo, allora, lasciatemi spendere un appello per un intervento immediato, per dare risposte ai bisogni concreti dei territori del Nord-Ovest del Paese colpiti dal maltempo. Su questo tema, in accordo con gli attori del territorio, avevo presentato un emendamento per l'Alessandrino. Ora è tutto il Piemonte ad aver bisogno di attenzione e risorse. I Presidenti di Piemonte e Liguria hanno chiesto lo stato d'emergenza: l'Esecutivo si affretti in questo senso. Avrei voluto che quest'Assemblea desse un segnale ai territori con l'approvazione del mio emendamento sull'Alessandrino; non è stato così e il continuo ricorso alla fiducia da parte del Governo ci impedisce di dare un segnale, almeno con l'approvazione di un ordine del giorno. Il decreto agosto contiene di tutto, ma in questo caso non tiene conto di quello che serve. L'attenzione politica, però, non può e non deve mancare e dunque mi appello ai colleghi affinché si creino le condizioni per non lasciare soli i territori, le famiglie e gli imprenditori.

Sottosegretario, onorevoli colleghi, in apertura di questo breve intervento, lasciatemi mandare un saluto e un abbraccio a tutte le famiglie e comunità delle valli Tanaro, Gesso, Vermenagna, Valsesia e Val Roya e delle altre valli e territori colpiti dalla recente

Su questo tema voglio ringraziare il presidente Conte per la sollecitudine con cui ha espresso la volontà di interventi immediati, che seguiremo e accompagneremo, perché i

Venendo al merito del lavoro odierno, credo abbiamo tutti la consapevolezza che il decreto-legge oggi alla nostra attenzione per la conversione - peraltro, dopo un lavorio importante da parte di tutti i colleghi e, in particolare, della Commissione bilancio - sia straordinariamente importante per aiutare il nostro Paese, in tutte le sue articolazioni, la nostra comunità civile ad affrontare questa stagione di emergenza causata dalla pandemia che ha colpito e che continua a colpire tutto il mondo e anche le nostre comunità, con morti, ammalati e limitazioni, e che continua a richiederci in modo forte di non abbassare la guardia. È un decreto-legge che segue i decreti cura, liquidità, semplificazioni, rilancio e che in qualche misura ne integra l'opera, prevedendo il proseguimento delle tutele per il mondo del lavoro e andando a coprire i settori che erano rimasti scoperti, mettendo in campo nuove misure per fronteggiare la domanda di salute in questa stagione straordinaria, da tutti i punti di vista, e per permettere alla nostra sanità di strutturarsi al meglio per farlo. Si predispongono nuove misure per le scuole e per l'universo istruzione in generale, chiamato ad una prova complessa dev'essere messo in condizione di gestirsi in una rinnovata ordinarietà, perché sono in gioco il presente e il futuro dei nostri figli. Sono previste nuove misure per sostenere il lavoro delle nostre Forze armate e di sicurezza sicurezza e gli enti locali, che sono stati e sono al momento un vero e proprio fronte in cui si gioca lo scontro di quest'emergenza, dal cui esito dipendono le condizioni in cui vivranno le nostre famiglie e la qualità e il contesto in cui opereranno le nostre imprese, in tutte le forme di vita organizzata, e, in generale, in cui si snoderà la vita civile, sociale ed economica delle nostre comunità. poi misure specifiche a sostegno proprio del nostro sistema economico: delle micro, piccole e medie imprese, in generale, ma soprattutto dei settori particolarmente colpiti, quali quelli turistico, della cultura, della ristorazione, dello spettacolo, fieristico, termale, dello sport, ma anche del comparto manifatturiero, della pesca e dell'agricoltura; misure di semplificazione e adeguamento ai nuovi comportamenti; limitazioni imposte dal perdurare dell'emergenza, come le regole che sovrintendono alla vita condominiale. contiene anche - o forse dovrei dire soprattutto - misure che orientano e incentivano a una vita e a uno sviluppo orientati in modo più sostenibile: basse emissioni, maggior recupero e riutilizzo e minore spreco di risorse nel campo delle costruzioni, dei materiali, della mobilità e dei trasporti; e poi infrastrutture, editoria e molti altri settori di intervento, nonché proroghe in campo fiscale: tutte misure per affrontare l'emergenza, ma anche orientate a quell'idea di stagione nuova che si aprirà davanti a noi all'uscita - speriamo presto - da quest'emergenza. fatto in Commissione ha ulteriormente completato e arricchito questo lavoro con chiarimenti normativi, implementazioni e affinamenti di norme già presenti nel decreto e in quelli precedenti, con il con il riconoscimento di situazioni particolari, quali quelle legate alla quarantena di componenti delle famiglie o delle persone in fragilità; nel caso della quarta gamma e delle colture colpite da gelate per il comparto agricolo, ha inserito ulteriori misure per gli enti locali; in agricoltura, per il comparto vitivinicolo; e poi, misure in campo fiscale. Tutto questo, ovviamente, è motivo di soddisfazione e gratitudine per il lavoro che, con la collaborazione di tutti, si è potuto fare nel clima giusto. Voglio per questo ringraziare i relatori, i rappresentanti di Governo e anche le opposizioni per il clima di collaborazione in cui si è potuto lavorare. Rimane il rammarico per ciò che non si è potuto fare e che necessariamente sarà rinviato alla legge di bilancio o ad altri provvedimenti: emendamenti come il 58.9, che puntava a chiarire le modalità di applicazione di una norma che è attuata in modo difforme in vari territori; al tema dei requisiti per la connessione all'attività agricola degli agriturismi (si mirava a introdurre linee guida nazionali che fossero applicate sui territori in modo uniforme dalle singole Regioni). a emendamenti che tendevano a cancellare strumenti e norme che non hanno più ragione di esistere, come il 103.4, che puntava ad abolire il contrassegno di Stato sugli alcolici: uno strumento che nasceva per controllare il versamento delle accise, ma che, ora che essa è assolta alla fonte, non ha più ragione di esistere; o che puntava a dare garanzia di qualità dei prodotti, ma che adesso, con il *packaging,* l'immagine delle imprese che producono questi prodotti e la comunicazione, non ha più alcuna ragione di esistere.

per la logistica, i magazzini, la contabilità e i controlli e crea enormi diseconomie alle imprese che devono tenere magazzini distinti per il mercato italiano e quello estero, con costi di magazzinaggio, contabilità, gestione e logistica. a emendamenti miranti a normare ambiti dell'attività umana, strumenti o materiali di nuova utilità e utilizzo, come nel caso del 58.0.48, volto a normare in modo puntuale l'utilizzo del digestato, cioè il risultato della digestione anaerobica delle biomasse, degli scarti e dei reflui agricolo-zootecnici; si tratta di una necessità importante per orientare in modo virtuoso la migliore qualità di questo prodotto, che può sostituire in larga parte il concime chimico e migliorare i reflui zootecnici restituiti al terreno, in ultima analisi migliorando la tessitura, la fertilità del terreno e il rapporto con le acque. si farebbe chiedendo maggiore qualità e controlli più rigidi agli operatori e, a fronte di ciò, permettendo un più ampio utilizzo. Voglio esprimere il rammarico per l'emendamento 11.0.2, che avrebbe permesso l'immediato utilizzo delle risorse destinate ai lavoratori colpiti da malattie conseguenti all'inalazione di fibre di amianto nel settore rotabile ferroviario. Alcuni di loro sono anche esodati, cioè senza lavoro, in attesa del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 208 del 2015, comma 277, che faceva riferimento ai benefici dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992.

può trarre da quest'emergenza una sfida forte e rinnovata per uscirne migliore. A noi sta il compito di fornire alle imprese, alle famiglie e ai cittadini gli strumenti per poterlo fare al meglio.

anch'io voglio iniziare questo intervento manifestando solidarietà ai territori e alle popolazioni colpite dai nubifragi che si sono riversati su Piemonte, Liguria, Lombardia e in generale sul nostro Paese. Lo faccio in quest'occasione, a maggior ragione, dopo le dichiarazioni di un rappresentante del Governo che, anziché esprimere giudizi, dovrebbe individuare soluzioni. Mi riferisco al ministro Costa che, dal caldo e comodo ufficio del suo Ministero, si è permesso di accusare coloro che sono primi cittadini non solo nel rappresentare una comunità, ma anche nell'affrontare l'emergenza, che in questi giorni, insieme alla propria comunità, stanno affrontando con le loro mani e con il loro impegno in prima persona il tentativo di risistemare ciò che il maltempo ha devastato. A loro va sicuramente il nostro rispetto, a prescindere dall'appartenenza politica, perché lo meritano. *(Applausi).* Oggi fare il sindaco significa cercare di dare risposte alle proprie comunità, senza mezzi, senza personale a volte, senza nemmeno le gratificazioni che derivano dal loro impegno. È vergognoso che un Ministro affermi che il dissesto idrogeologico non è mai stato affrontato non per carenza di fondi, ma per le carenze dei Comuni. Se un Ministro di questo genere ha diritto di rappresentare il nostro Paese, credo che siamo scaduti a livelli bassissimi. È lo stesso Ministro che, in tutti i provvedimenti che abbiamo portato avanti anche in questi mesi, è stato sempre il "signor no": il "signor no": no ad ogni tentativo, anche del nostro movimento, di apportare modifiche correttive a un sistema assolutamente ingessato; no, anche in questo decreto, alla richiesta di stanziare 100 milioni - cifra che ritenevamo ragionevole, in un provvedimento che stanzia 25 miliardi - per dare le prime risposte al dissesto idrogeologico. Noi l'abbiamo fatto: abbiamo presentato un emendamento, lo abbiamo discusso con la maggioranza e col Governo, ma la risposta è stata: no, ci sono altre priorità. Stiamo vedendo - ahimè - anche in queste ore che è una priorità del nostro Paese e voi non la state affrontando minimamente. Intervengo senza grande entusiasmo rispetto a questo provvedimento, perché è il quinto dell'attuale fase emergenziale,

in un certo senso, è calmierata dallo stanziamento di questi 100 miliardi che avete versato nella nella spesa pubblica, ma che affrontano solo in via emergenziale la cassa integrazione con sussidi, indennità, contributi e *bonus* che non risolvono assolutamente il problema che sta vivendo il nostro Paese. I problemi che state gestendo si ripeteranno e si manifesteranno in tutta la loro drammaticità quando queste risorse finiranno (e, prima o poi, questi stanziamenti finiranno). Avete speso 100 miliardi avete intenzione di spenderne altri 200 l'anno prossimo con il *recovery fund*, ma va ricordato che tutte queste risorse sono a debito, non sono nelle disponibilità del nostro sistema produttivo. Vi indebitate ed è opportuno farlo, ma se ci sono soluzioni strutturali, non forme di sussidi e indennità che lasciano il tempo che trovano e rinviano il baratro verso il quale stiamo andando. È qui che si rispecchia la differenza di mentalità tra la vostra parte politica, che è quella della sinistra e dei 5 Stelle, che almeno dal punto di vista economico hanno la stessa visione, e la nostra parte. Riteniamo evidente che tutte queste forme di sussidio e di indennità e di indennità siano finanziate o a debito o con la raccolta delle tasse. Abbiamo una visione diversa: no a indennità, no a sussidi, no a redditi di cittadinanza o di emergenza. Lasciamo i soldi nelle tasche delle famiglie, degli imprenditori, dei commercianti e degli artigiani, perché possano lavorare e dare posti di lavoro. *(Applausi).* In questo modo si potrà avere una società sana, costruita sul lavoro non su sussidi o su forme emergenziali come quelle che proponete. Avete una visione dell'economia assolutamente distorta e pensate che il nostro Paese possa vivere con questi strumenti, ma è evidente che prima o poi il castello crollerà. Ci troviamo ormai in una situazione in cui la barca fa acqua da tutte le parti e continuate a mettere toppe a destra e a manca, in varie direzioni, senza trovare le soluzioni definitive. Bisogna alleggerire il carico, che è fatto di tasse e burocrazia. Sono stati approvati, in questi tre anni, due decreti-legge che dovevano semplificare il mondo degli appalti, il nostro Governo, sicuramente ostacolati da una visione dei 5 Stelle, che non era la nostra, e infatti quel decreto-legge non ha raggiunto tutti gli obiettivi che doveva, e con un decreto semplificazioni che allo stesso modo non ha semplificato assolutamente nulla.

e la burocrazia serve, perché tendenzialmente siamo tutti disonesti e quindi, per impedire che i disonesti facciano quello che vogliono, ci vogliono regole infinite, impossibili da gestire e da affrontare per chi lavora. Alla fine raggiungete solo un obiettivo: chi è disonesto lo rimane, riesce a evadere e ad evitare la burocrazia e fa quello che vuole, nonostante tutti i vostri lacci e lacciuoli. Registro anche che, dalla Nota di aggiornamento al DEF che avete da poco sfornato, si presume ancora adesso di poter raccogliere ingenti risorse dalla lotta all'evasione fiscale: l'ennesima fantasia; l'ennesima follia. D'altra parte, non vi accorgete che, col carico fiscale enorme, fate chiudere le aziende e le attività artigianali e commerciali e fate sì che quelli che erano lavoratori oggi diventino disoccupati che hanno bisogno di sussidi, cassa integrazione e redditi di cittadinanza. Con la burocrazia mettete fuori gioco gli onesti, che vogliono e si trovano costretti ad adempiere a tutte queste forme di vincoli da parte dello Stato e fate sopravvivere chi invece riesce ad evitare con la disonestà tutte queste procedure. Questo è il modello di società vostro, che sicuramente porterà al fallimento di uno dei sistemi economici più all'avanguardia del nostro Paese. Questo è il dramma che stiamo vivendo, nel totale silenzio e nell'indifferenza: in una situazione surreale, qui non ci stiamo accorgendo che, finiti i 100 miliardi e finiti i 200 del avremo solo più debito pubblico, senza aver minimamente affrontato la sfida di cambiare la pressione fiscale e il carico burocratico che oggi più che in passato dovevamo affrontare. Avevamo un'occasione storica, con tutte le risorse che l'Europa generosamente ci ha autorizzato a utilizzare a debito, ma non lo stiamo facendo. L'occasione la stiamo perdendo per colpa vostra. Per l'ennesima volta caricate cittadini e lavoratori di burocrazia e tasse e condannate tutti noi a un inesorabile declino. Speriamo che finisca questo periodo, ma il rischio è di raccogliere solo le ceneri. *(Applausi)*.

Signor Presidente, ancora una volta siamo chiamati a convertire un decreto-legge in tutta fretta e in un clima di apprensione. Spesso, quando trascorriamo le giornate qua, all'interno dei locali del Senato, ci sembra quasi che la pandemia sia un po' lontana da queste sale. Invece, la scorsa settimana è entrata nel palazzo del Senato e ha contagiato due colleghi: Marco Croatti e Francesco Mollame, a cui ovviamente vanno il nostro abbraccio e un augurio di pronta guarigione.

La mancata conversione avrebbe significato: la mancata proroga della cassa integrazione, con migliaia di imprese costrette a licenziare nell'immediato i propri dipendenti; la mancata proroga del pagamento delle imposte sui redditi e dell'esonero da TOSAP e COSAP per bar e ristoranti; la mancata proroga degli ammortizzatori sociali Naspi e della disoccupazione per i collaboratori. I lavoratori dipendenti stagionali del turismo non avrebbero potuto ricevere l'indennità di 1.000 euro prevista dal decreto i lavoratori marittimi avrebbero visto decadere il diritto all'indennità di 600 euro per i mesi di giugno e luglio. Ancora, non ci sarebbe stato l'aumento da 600 a 1.000 euro delle indennità per il mese di maggio in favore dei liberi professionisti iscritti a enti di previdenza obbligatoria, così come il così come il sussidio di 600 euro per i lavoratori sportivi. Non ci sarebbe stata la conversione della misura della decontribuzione del 30 per cento per le assunzioni nelle Regioni del Sud. Non ci sarebbe stato neanche l'incremento della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali: 1,6 miliardi di euro in più per compensare Comuni, Province e città metropolitane dalla perdita di entrate locali conseguenti al Covid.

Oggi abbiamo sentito alcune considerazioni da parte dei colleghi dell'opposizione. Qualcuno, credo il senatore Urso, ha chiamato il decreto agosto un "polpettone senza significato". Credo che anche tanti colleghi di opposizione Credo che anche tanti colleghi di opposizione oggi sappiano quali sarebbero state le gravi conseguenze in caso di mancata conversione di questo decreto-legge credo che si sarebbero dovuti preoccupare del fatto che 83 emendamenti che sono stati approvati, proposti dall'opposizione, non sarebbero stati convertiti insieme ad esso. Per consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali causate dal Covid-19 sono state impiegate dal Governo Conte risorse per 100 miliardi di euro, 25 dei quali stanziati nel solo decreto agosto che siamo chiamati a convertire. Sappiamo che da questo *shock*, da questa emergenza potremmo trarre un'occasione unica, da non perdere, per mettere in discussione tutti quegli aspetti della vita del Paese che hanno condizionato negativamente il progresso economico e sociale negli ultimi vent'anni. Sappiamo tutti delle grandi opportunità che potremmo trarre dalle risorse che verranno reperite con il programma *next generation* *EU*, che prevede di raccogliere sui mercati fondi per 750 miliardi di euro, dei quali circa 191 (209, (209, se consideriamo anche altri fondi di minore entità) saranno destinati all'Italia, 80 dei quali a fondo perduto. Per la prima volta, quello che potrebbe diventare un fondo sovrano europeo, alimentato con l'emissione di titoli europei di debito, sovvenzionerà i singoli Stati membri con trasferimenti a fondo perduto, esattamente come fa lo Stato italiano nei confronti delle proprie Regioni. Inaspettatamente, sicuramente a causa di una grave situazione di emergenza, abbiamo fatto un balzo enorme nell'integrazione europea e ora siamo chiamati a spendere, e a spendere bene, le risorse che dovranno arrivare. Il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni Silveri, poche settimane fa, ci ha confermato che le risorse del *recovery fund* non possono essere usate per ridurre la pressione fiscale. Credo però che potranno essere usate per innovare il nostro sistema fiscale, per sviluppare nuovi strumenti tecnologici che rendano più facile la vita dei contribuenti e meno conveniente evadere le tasse. Non esiste solo un problema di carico fiscale eccessivo sui redditi medio-bassi. Sappiamo che tra i 28.000 e i 40.000 euro di reddito l'aliquota marginale media, cioè quello che prende il fisco su ogni euro addizionale guadagnato, varia dal 45 al 60 Il problema esiste, è grave, ma non è certo l'unico. Il nostro fisco è quasi imperscrutabile, è ignoto. Da questo scaturisce la paura dell'ignoto e il nostro sistema impositivo fa paura, soprattutto alle imprese che vorrebbero esercitare attività economica, economica, investire e innovare. Occorre - e per questo mi rivolgo anche al Governo - abbandonare i vecchi schemi di ragionamento sul fisco. Le disquisizioni sulle aliquote, di cui sentiamo parlare anche in questi giorni, sono utili, sicuramente poco appassionanti e spesso rischiano di essere vane. È necessario invece coinvolgere nella riforma del sistema fiscale soggetti che siano in grado di realizzare infrastrutture complesse, che rendano semplice il calcolo e il pagamento delle tasse. Il contribuente, il piccolo imprenditore e il professionista, che sono l'ossatura del nostro sistema economico, devono essere in grado di sapere in modo semplice e immediato, prima di accettare un nuovo incarico e di realizzare una nuova opera, quante tasse in più dovranno pagare in corrispondenza di un determinato maggiore ricavo. Chi esercita un'attività economica dev'essere liberato dagli adempimenti fiscali, dalla burocrazia fiscale. Il livello tecnologico raggiunto è tale da poter pensare ad un sistema di prelievo o micro prelievo immediato, che liberi la piccola impresa o il professionista da qualsiasi ulteriore o successivo onere o adempimento fiscale. Il lavoratore autonomo in questo dev'essere parificato a quello dipendente. Deve avere lo stesso diritto di non vivere nella preoccupazione di adempimenti o controlli fiscali futuri e deve pensare solo a far crescere la propria impresa. Solo così potremo avere certezza nel rapporto tributario. La complessità e l'incertezza forse sono tra le maggiori cause dell'evasione fiscale, ancora di più della quantità o dell'entità delle aliquote, che è l'argomento di cui si dibatte in questi giorni. Chi esercita un'attività economica spesso vive nel terrore di vedersi recapitare pretese che non aveva previsto. Questa condizione contribuisce a creare un clima di paura, che disincentiva e svilisce investimenti e iniziative imprenditoriali. Con i soldi del *recovery fund* non possiamo ridurre la pressione fiscale, come ci dice il commissario europeo agli affari economici, però possiamo usare i fondi per rendere più semplice e più trasparente il rapporto tributario. La tecnologia può e deve essere utilizzata anche per rendere più facilmente fruibili gli incentivi fiscali. Per quanto riguarda il superbonus, voglio ricordare innanzitutto ai colleghi del nostro Gruppo che è una misura del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo introdotto per la prima volta la possibilità di cedere senza limiti i crediti derivanti dalle detrazioni per efficientamento energetico. Attraverso l'uso della tecnologia, possiamo pensare di rendere più fluida la circolazione di questi crediti fiscali. Perché, una volta certificati attraverso un portale come il cassetto fiscale, non si può pensare di consentire l'utilizzo di questi crediti anche quale corrispettivo per l'acquisto di beni e servizi? Ci sono dei vincoli, Ci sono dei vincoli, però credo che la tecnologia sia tale da poterne tenere conto nella circolazione dei crediti. D'altronde, dal punto di vista normativo, in realtà, i crediti nei confronti dello Stato possono essere ceduti a terzi dal 1923, da da quando è entrato in vigore il regio decreto n. 2440. Si può fare, quindi, e nel frattempo abbiamo anche raggiunto un livello di tecnologia che ci consente di farlo anche in modo più fluido e sicuro. Da un articolo apparso il 24 settembre sul «Corriere della Sera», che raccontava di uno scontro tra il Garante della *privacy* irlandese e il colosso Facebook, emerso che il valore economico stimato dei dati personali dei cittadini europei che ogni anno vengono trasferiti verso gli Stati Uniti e che vengono utilizzati da Facebook come fosse materia prima è pari a 7.000 miliardi di euro annui. personali che cediamo ogni anno e che valgono 7.000 miliardi di euro vengono sfruttati economicamente e gratuitamente da imprese che li usano per produrre servizi e per conseguire legittimamente ricavi in tutto il mondo. Si possono utilizzare le risorse del *recovery* per realizzare un sistema che sia in grado di intercettare e tracciare questi dati. Si può prevedere una forma di ristoro nei confronti dei loro legittimi proprietari, ovvero nei nostri confronti. Temiamo magari una guerra commerciale e forse abbiamo qualche remora su questo, però il problema va affrontato con ragionevolezza, la stessa che deve impedirci di sperperare un patrimonio di 7.000 miliardi di euro. Signor Presidente, con l'approvazione di questo decreto-legge si conferma la volontà di sostenere con uno sforzo senza precedenti le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane, proteggendole dalle conseguenze economiche negative generate dall'emergenza epidemiologica.

la visibilità mediatica anche con idee la cui portata potrebbe non essere compresa nell'immediato dall'elettorato; però, dobbiamo farlo: dobbiamo programmare il futuro del Paese. *(Applausi).*

Signor Presidente, faccio alcune brevi considerazioni anche rispetto all'andamento del dibattito e alle questioni che diversi colleghi senatori hanno posto all'attenzione del nostro confronto. La prima è relativa al percorso che abbiamo seguito. Continuo a pensare che l'accusa che ci viene rivolta rispetto all'utilizzo del voto di fiducia, a detta di alcuni improprio, non tiene conto, a mio avviso, del lavoro prezioso e importante che abbiamo svolto in Commissione. Abbiamo votato gli emendamenti, abbiamo realizzato un confronto politico che considero serio e produttivo, anche con le forze di opposizione; abbiamo convertito questo decreto-legge anche grazie a una collaborazione preziosa con il Governo,

Abbiamo affrontato temi importanti, che credo siano un elemento prezioso per la nostra democrazia, per il confronto politico tra

Rispetto agli altri passaggi parlamentari di conversione, dal decreto-legge cura Italia fino al decreto rilancio, noi consideriamo questo percorso particolarmente importante, anche per effetto di un confronto costruttivo. modo, definire le proposte della maggioranza e del Governo senza un'identità, una visione, io continuo a pensare che sia un elemento di debolezza, perché l'identità e la visione ci sono all'interno dei nostri progetti e delle proposte con le quali questo Governo ha inteso portare via l'Italia dalla crisi pandemica. C'è un'identità quando parliamo di lavoro; c'è un'identità quando parliamo di sostegno alle imprese; c'è un'identità quando parliamo di sostegno alle famiglie; c'è un'identità quando, attraverso interventi specifici, abbiamo messo Regioni ed Enti locali nelle condizioni di collaborare con lo Stato per uscire da questa crisi. Non mi si può dire che non c'è una visione, perché il progetto che il Governo ha messo in campo per attraversare e uscire da questa crisi poggia su dei valori precisi di non lasciare indietro le persone e contemporaneamente di unire e non dividere il lavoro dal capitale, il lavoro dall'impresa. Non c'è nessuna ideologia retroattiva nel considerare l'impresa preziosa per il sistema territoriale; non abbiamo nessuna dietrologia ideologica e non consideriamo le partite IVA, i lavoratori autonomi come elementi di evasione fiscale; li consideriamo elementi fondamentali di una comunità, perché questo è l'indirizzo politico contenuto all'interno di tutti i provvedimenti che abbiamo determinato per attraversare questa crisi. sia nelle procedure sia nel merito, attraversare un'emergenza così grave, che non ha colpito solo l'Italia ma che ha colpito al cuore il mondo nella sua interezza, ovviamente ha richiesto anche l'utilizzo di procedure in emergenza, perché siamo all'interno di un'emergenza. Non è solo un problema di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; siamo all'interno di un'emergenza perché le dinamiche pandemiche hanno prodotto uno *shock* economico rilevantissimo. Quando si perdono oltre 10 punti di PIL è inevitabile che siamo dentro uno stravolgimento delle dinamiche economiche e sociali che richiedono azioni strutturali. decreto agosto è un ponte verso l'utilizzo del nuovo volto che l'Europa metterà a disposizione per superare questa crisi e costruire un nuovo modello di sviluppo economico; è un modello di sviluppo economico che appoggerà su un'economia ambientalmente sostenibile, su un'Italia più digitale, sull'innovazione e sulla ricerca indispensabili da accompagnare ad una nuova idea dello sviluppo economico. È un cambiamento, perché non si riparte con gli strumenti del passato; si devono individuare nuove dimensioni economiche e sociali indispensabili per favorire lavoro e crescita economica. Sarà una nuova crescita economica, non uguale a quella ante crisi pandemica. Ne stanno discutendo in ogni angolo del globo e dunque anche all'interno dell'Europa, per questo lo definisco il ponte verso la dinamica europea e per questo mi sembra ingeneroso e non giusto accusare la maggioranza e il Governo di non disporre di una visione. visione. Con altrettanta chiarezza dico che per noi gli ammortizzatori sociali non sono una forma di intervento assistenziale. La loro selettività è fondamentale per salvare le imprese; è decisiva per mettere in sicurezza pezzi del nostro tessuto produttivo. Come si fa a definire un ammortizzatore sociale un intervento assistenziale? Se collochiamo il lavoro e l'impresa in una forma di assistenzialismo, è l'identità precisa di un Paese che decide di costruire le condizioni fondamentali per proteggere il lavoro, salvare le imprese e contribuire, anche attraverso un nuovo impegno dello Stato, ad nuova riconversione economica di pezzi della nostra economia, certamente più orientati verso la sostenibilità ambientale. *Green economy* significa questo: economia circolare, circolare, innovazione e ricerca; sono punti di contatto che sono parte integrante del progetto politico di questa maggioranza. Per questo dico che c'è una visione, un'identità. Certamente stiamo attraversando un'emergenza, ma c'è un'idea della società sulla quale noi abbiamo costruito la nostra risposta alla crisi pandemica. Ancora, sono diverse le misure che abbiamo introdotto anche sul versante economico; non abbiamo avuto il tempo di valorizzarle, ma considero molti interventi positivi quali, ad esempio, quelli adottati nei confronti delle imprese. La sospensione temporanea degli ammortamenti, per quello che riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali, avrà un effetto positivo, cioè proteggerà diverse piccole e medie imprese dalla loro possibile estensione verso le procedure difficili che la norma relativa alle procedure fallimentari determina. Si sta facendo ogni azione per mettere in sicurezza un numero rilevante di imprese, per poter ripartire, per poter costruire un'idea di futuro del nostro Paese. gli interventi che abbiamo adottato nei confronti della piccola e media impresa, del lavoratore autonomo, delle partite IVA. Probabilmente non saranno completi, non si concluderanno certamente all'interno di questi provvedimenti perché abbiamo bisogno di riposizionare ovviamente lo Stato dentro le dinamiche delle infrastrutture, dell'economia, del sistema infrastrutturale anche digitale che dobbiamo contribuire a realizzare. Non sono gli unici interventi; non si possono definire mance né *bonus* a *go go*. Sono interventi fondamentali che hanno un proprio profilo e un loro orientamento, e che credo aiuteranno questo Paese a uscire dalla crisi, ma appoggeranno questa crisi su una nuova visione dell'economia e della società. Colleghi, ho cercato di rappresentare taluni elementi in questa mia replica, certamente non per accusare qualcuno, ma semplicemente per ritenere quella che abbiamo compiuto nella conversione del decreto-legge una scelta coerente con una visione e un'identità che ci accomunano. Una visione e un'identità che hanno deciso di lavorare per allargare l'area dei diritti, perché utilizzare oltre 300 milioni di euro per dare garanzie a un lavoratore immunodepresso o a un cittadino che sta subendo cure oncologiche è secondo me dovere di un Paese; un dovere del sistema pubblico. Garantire e allargare l'area dei diritti è un qualcosa che ci appartiene. Restituire centralità al lavoro è una scelta culturale e politica che ci vede uniti in un'idea di futuro del nostro Paese. Saldare il capitale con il lavoro e toglierci dalle contrapposizioni ideologiche del passato è l'elemento fondamentale di un'idea di futuro dell'economia e della società. Cominciamo a lasciare al passato il dibattito del passato e cerchiamo di contribuire insieme alla costruzione e alla lettura di una nuova dimensione sociale ed economica. la politica torna a essere credibile, le istituzioni tornano a essere fondamentali per garantire interventi indispensabili alle famiglie e alle imprese. Ho fatto il sindaco e ho sentito parlare in maniera non appropriata delle dichiarazioni del ministro Costa. Non penso che il Ministro avesse alcuna intenzione di scaricare sui Comuni un tema che non si può imputare alla responsabilità del Ministro. Quello che è successo in Piemonte è una grave calamità; è una tragedia per quel territorio. Occorre intervenire, ma non dobbiamo dimenticare che le ragioni le ragioni del blocco del Patto di stabilità, le ragioni del blocco degli investimenti degli Enti locali hanno radici lontane: risalgono alla stagione dell'*austerity*; risalgono al volto di un'Europa diversa rispetto a quello che stiamo costruendo costruendo e con il quale stiamo contribuendo a dare al perimetro europeo una nuova visione. Cominciamo ad abbandonare queste idee perché non c'è dubbio che l'assetto idrogeologico del nostro territorio e i suoi interventi di manutenzione richiedono una quantità di investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto al passato; ma i Comuni non erano nelle condizioni di investire perché, purtroppo, per tanti anni tutto il sistema pubblico è stato costretto, attraverso il Patto di stabilità interno, a non poter sviluppare gli investimenti. Per aggredire la crisi del 2008 siamo stati costretti a rinunciare agli investimenti e i Comuni hanno ridotto la manutenzione del territorio, e dunque oggi dobbiamo rimettere in cammino gli investimenti. Questo Paese ripartirà dagli investimenti, non ci sarà nessuno spazio per ripartire senza gli investimenti degli Enti locali e senza un nuovo perimetro, una nuova individuazione del ruolo della pubblica amministrazione. Dobbiamo dare corso a queste azioni, perché se vogliamo ripartire con gli investimenti dobbiamo ristrutturare le nostre stazioni appaltanti, dobbiamo creare ambiti territoriali ottimali, dobbiamo ricostruire il volto del sistema socio-sanitario nel territorio. Ecco che ripartire con gli investimenti e anche ripartire con un piano straordinario di riassetto idrogeologico del nostro Paese è una priorità: nessun conflitto, nessun capo di imputazione nei confronti del Ministro, nessuna accusa nei confronti dei sindaci. A noi spetta il compito di rammendare, di mantenere, di rimettere al centro gli investimenti, per realizzare un grande piano di contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro Paese. Queste sono le azioni

proposte dalla Commissione in sede referente, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

una nuova finestra") Onorevoli colleghi, la Presidenza ha valutato, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter* del Regolamento, l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del decreto-legge n. 104, recante sostegno e rilancio dell'economia. La Presidenza dichiara improponibili le disposizioni del maxiemendamento presentato dal Governo che riproducono il contenuto dei seguenti emendamenti approvati in sede referente: 30.0.4, limitatamente agli ultimi due periodi; 32.22; 42.0.1; 44.0.3; 44.0.4; 54.0.1; 77.37, limitatamente al comma 2-*quater*; 77.62, limitatamente al comma 3-*bis*; 82.0.3; 100.10, limitatamente ai commi da 10-*ter* a 10-*septies*; 112.0.5. I seguenti emendamenti confluiti nel maxiemendamento sono ammissibili a condizione che vengano ricollocati come di seguito indicato: 47.2 all'articolo 51; 058.1 all'articolo 60; 59.0.13 all'articolo 60;

51; 96.0.7 all'articolo 51; 96.0.24 all'articolo 51; 109.1 all'articolo 64. Ha chiesto nuovamente di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà. onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1925, nel testo ritenuto proponibile dalla Presidenza,

come modificato dal Governo. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della questione di fiducia preannunciata dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge sostegno e rilancio dell'economia. Per la discussione, che avrà inizio domattina alle ore 9,30, sono stati ripartiti dieci minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama. Il calendario è integrato domani, alle ore 12,30, con le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. Sono state ripartite tra i Gruppi tre ore comprensive di interventi nella discussione e dichiarazioni di voto sulle eventuali risoluzioni presentate. Martedì 13 ottobre, alle ore 15,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020. **Atti